Non siamo riusciti a votare ancora gli emendamenti; abbiamo concluso ieri la fase di espressione dei pareri sugli emendamenti depositati da tutte le forze politiche manca ancora il parere su una mole di emendamenti e subemendamenti cospicua (mi riferisco agli ultimi emendamenti depositati dal Governo e dal relatore e ai subemendamenti agli stessi).

senatrice De Petris)*.

votazione ed è quindi evidente, Presidente, che noi non possiamo far altro, a questo punto, che chiedere urgentemente la riunione dei Capigruppo. Mi lasci dire almeno che noi avevamo fatto delle richieste precise, che qui in Aula

Signor Presidente, per ora mi limito a confermare, anche da parte del Partito Democratico, la richiesta della convocazione immediata della Conferenza dei Capigruppo, perché non c'è davvero limite all'incredibile, in questi lavori. Penso che il presidente Pesco sarebbe dovuto arrivare in Aula oggi, dopo tutto il pregresso, dicendo semplicemente che avevano scelto, come Commissione, di venire in Aula senza relatore. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Penso che sia veramente scandaloso che, dopo quanto accaduto in questi giorni, si arrivi a rimettere alla Presidenza la scelta di come procedere, di fronte all'unica alternativa, che è quella di lavorare ancora per alcuni giorni, soprattutto perché - caso mai visto - non si è fatto ancora un voto sul disegno di legge di bilancio.

per tutte le motivazioni dianzi esposte e per molte altre ancora, che nascono da quindici giorni a partire da ora e da una Commissione che, fino adesso, non ha, su questa manovra invisibile, ancora espresso nemmeno un voto e la sta portando in Aula con un inedito assoluto nella storia della Repubblica italiana. Non siamo qui solo per stigmatizzare una iconoclastia, una rottura totale della Costituzione,

che cosa fare e cerchiamo di capire com'è possibile, se è possibile, quando è possibile, leggere il contenuto fantasma di questa manovra fantasma.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio. Nella seduta di stasera, che si concluderà alle ore 24, avrà inizio la discussione generale. Tale discussione riprenderà nella seduta di domani, dalle ore 9 alle ore 12. A tal fine sono state ripartite otto ore. Conclusa la predetta fase procedurale, si passerà al voto degli emendamenti e degli articoli della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, secondo quanto stabilito dall'articolo 129 del Regolamento. Successivamente, si esaminerà la prima sezione del disegno di legge, che consta di un solo articolo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 20. Poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sulla prima sezione del disegno di legge, la Conferenza dei Capigruppo ha già previsto in linea di massima l'articolazione dei tempi successivi, cosicché la discussione sulla fiducia avrà la durata di circa quattro ore, in base a specifiche richieste dei Gruppi. È stato altresì stabilito che alle ore 22 di domani, con ripresa diretta televisiva, si svolgeranno in un'unica fase le dichiarazioni di voto sulla fiducia e sul complesso della legge. Seguirà la chiama. Una volta votato l'articolo 1 della prima sezione, la seduta dovrà essere sospesa per consentire al Governo di presentare la seconda Nota di variazioni al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla 5ª Commissione permanente. L'Assemblea procederà quindi al voto della Nota di variazioni e al voto finale del disegno di legge, con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo, a nome del Gruppo Forza Italia, abbiamo presentato proposte di calendario alternative. Come abbiamo spiegato ai colleghi e come vogliamo comunicare all'Assemblea, riteniamo che sia un'eccentricità assolutamente inaccettabile - e usiamo ovviamente un'espressione blanda, riservandoci in altre sedi di essere molto meno blandi

votato in Commissione, una Commissione che è stata riunita permanentemente per quindici giorni con commissari bilancisti segregati a parlare del nulla. Noi - come ha detto il presidente Calderoli - dovremmo discutere del nulla, nel senso che dovremmo fare una discussione su argomenti a piacere da adesso a mezzogiorno di domani, dal momento che il contenuto della manovra non è quello del

Domani arriverà il maxiemendamento. La nostra proposta è articolata su due punti: il primo punto è che si abbia il coraggio di metterci la faccia e si torni qui tutti il 24 e il 26 dicembre. Rimandiamo la manovra in Commissione immediatamente e votiamo articolo per articolo tutti gli articoli segnalati. Cerchiamo di fare una figura civile nei confronti del Paese e dei nostri rappresentati: tutti qui il 24 e il 26 dicembre. Misto-LeU)*. Il Governo sembra invece intenzionato a trascorrere le vacanze a casa, circondato dall'affetto dei suoi cari. Questo naturalmente fa piacere anche a noi, ma stiamo parlando della manovra di bilancio che deciderà i destini del Paese e li cambierà in peggio, molto in peggio. In estremo subordine, chiediamo quantomeno di essere messi nella condizione di parlare e, quindi, di non comprimere i tempi del dibattito come faremo domani con la diretta televisiva alle ore 22, in concorrenza con Marzullo o con Consorzio Nettuno. *(Applausi

in un ravvedimento operoso e attivo del Governo, se non per noi, quantomeno per gli italiani che stanno continuando a illudere con *slogan* senza contenuti.

che in Commissione bilancio non si tenesse neanche una votazione; gli esperti della Commissione bilancio lo sanno bene: neanche una bocciatura tecnica degli emendamenti

che non sono stati neanche presentati dai singoli in Commissione. Questo per farvi capire che siamo arrivati, ormai, all'esproprio totale, e non solo del Senato, perché la Camera ha votato una manovra manovra che non esiste, sulla quale, tra l'altro, noi adesso dovremmo iniziare la discussione generale. Abbiamo tentato con garbo - che dobbiamo fare? - di far comprendere che è

Governo di dire qualcosa, che cosa ne pensasse, se c'era la possibilità di lavorare su alcuni temi e di dare anche il nostro contributo. Siamo stati messi nella condizione di non poter lavorare. Dico anche di più. In realtà,

della Commissione bilancio, che non si voleva assolutamente svolgere alcun tipo di lavoro all'interno della Commissione. Per questo non è stato espresso nessun voto, per questo non è stata fatta neanche una votazione; l'esito doveva essere quello: arrivare in Assemblea al buio, senza relatore. Questo è quello che voi pensate che sia - e come debba essere ridotta - la democrazia parlamentare! Siccome il presidente Calderoli è relatore di una proposta di legge di revisione costituzionale, io vi dico di andare anche oltre: assumetevi la responsabilità, e su questo discutiamo, che

quello che dovete bocciare, bocciatelo, quello che dovete approvare, anche i vostri emendamenti, approvateli. Almeno saranno chiari i contorni degli emendamenti che volete approvare. Cerchiamo, in qualche modo, di riportare i lavori su un binario di ordinarietà. I tempi ci sono. Si può tornare in Commissione. Siamo ancora lontani dalla vigilia e da Natale. Abbiamo tutta la possibilità, finalmente, di farlo. E lo dico anche a a tutti i senatori di maggioranza: questo non è un problema solo delle opposizioni, ma è un problema di dignità del Parlamento. Riprendiamo in mano la possibilità di conoscere, di agire, di poter esercitare pienamente il nostro mandato.

Nessuno di noi vuole l'esercizio provvisorio; assumiamoci però la responsabilità di ritornare finalmente a dare una possibilità a

di leggi di bilancio, di discussioni in Commissione, ma mai - e sottolineo mai - mi era capitato di passare sei giorni e sei notti senza discutere né votare un emendamento, né della maggioranza, né dell'opposizione. Non un voto, signor Presidente. Una situazione senza precedenti, una mortificazione del ruolo che la Costituzione e i Regolamenti parlamentari affidano alla Commissione bilancio e al Parlamento della Repubblica. Sei giorni fino al paradosso di ieri sera, quando, alle ore 21,30, dopo un'infinita attesa e dopo una fiera delle ipocrisie, il Governo ha presentato queste paginette

per 10 miliardi di euro nel 2019, per 12 miliardi di euro nel 2020, per 16 miliardi di euro nel 2021, tagli alle pensioni, clausole di salvaguardia IVA: c'è un altro mondo, signor Presidente, c'è un'altra manovra, c'è un'altra legge di bilancio, che il Parlamento ha il diritto di discutere, avendo tutte le informazioni. Signor Presidente, questo Governo si definisce un Governo sovranista che dovrebbe tutelare le prerogative dell'Italia. Voi avete dato a Bruxelles, con il cappello in mano, numeri e tabelle che il Parlamento non ha: noi non abbiamo le informazioni che avete mandato a Pierre Moscovici, a Jean Claude Juncker e a Valdis Dombrovskis. Il Parlamento italiano ieri ha avuto cinque paginette - dico cinque - lette dal sottosegretario Castelli, che poco o nulla dicono su quanto questi emendamenti impattino sul prodotto interno lordo, sull'occupazione e sulla vita degli italiani, che vedranno tagliate le pensioni, aumentata l'IVA e realizzate cose molto diverse da quelle che avete promesso da ottantatré giorni a questa parte. Se le cose stanno così, signor Presidente, chiediamo a quest'Assemblea di difendere le prerogative del Parlamento, di tornare in Commissione e noi siamo disponibili a lavorare anche il 24 e il 26 dicembre per fare il nostro lavoro e il nostro dovere, che è quello di discutere con cognizione di causa questa manovra. Non stiamo parlando infatti di noccioline; stiamo parlando di miliardi di euro che cambieranno la vita degli italiani, spesso in peggio, e allora il Parlamento ha il diritto e il dovere di fare il proprio mestiere. Torniamo in Commissione. Dateci le informazioni che è nostro diritto avere; permetteteci di audire l'Ufficio parlamentare di bilancio, che non aveva validato le previsioni iperottimistiche della Nota di aggiornamento e che noi abbiamo il dovere di sentire per capire se i nuovi numeri macroeconomici che abbiamo letto sui giornali stanno in piedi, hanno senso oppure sono per l'ennesima volta campati in aria. Signor Presidente, glielo chiediamo con grande forza. Noi oggi abbiamo abbandonato per protesta, come gesto estremo, i lavori della Commissione bilancio. Non abbiamo fatto ostruzionismo in questi giorni. Abbiamo sempre tentato di lavorare con spirito costruttivo. Noi non le chiediamo altro che di avere la possibilità di fare il nostro lavoro, di discutere, di votare, di dare al Paese una decisione che avvenga su numeri, su fatti concreti, con cognizione di causa. Noi siamo chiamati a deliberare, ma per deliberare dobbiamo conoscere e noi oggi non conosciamo tutto ciò che dobbiamo sapere. Abbiamo il diritto e il dovere di farlo. A lei, Presidente, chiediamo di tutelare le prerogative del Senato della Repubblica.

Vice Presidenti. Grosso modo si è cercato di incanalare il dibattito su una concreta possibilità di interventi per tutti. Premetto che il capogruppo di Fratelli d'Italia, senatore Luca Ciriani, a nome di tutti noi si è dichiarato non solo disponibile, ma anche pronto a dare l'assenso a qualunque calendario ci consenta di fare un buon lavoro (che si tratti di lavorare il sabato, la domenica, il lunedì o quant'altro). Non credo, quindi, che nessuno

è arrivare all'esercizio provvisorio. La nostra opposizione patriottica, pronta a discutere in qualunque ora e in qualunque giorno, si ferma, non a parole ma nei fatti, di fronte all'eventuale pericolo di andare a un esercizio provvisorio che sarebbe estremamente dannoso, non per un Governo o per una maggioranza, ma per l'Italia. Qualunque sia il calendario, quindi, si tenga conto che dopo di noi di bilancio dovrà tornare alla Camera e non possiamo, in nessun caso, non tenere conto di una proiezione dei tempi che metta al sicuro l'approvazione della pessima finanziaria prima che scatti l'esercizio provvisorio.

*(PD)*. Signor Presidente, come dicevo poc'anzi, gli emendamenti presentati ieri dal Governo stravolgono completamente l'impianto della manovra,

nei pochi numeri che danno al Parlamento, ci dicono per esempio che la crescita, programmata inizialmente all'1,5 per cento, l'anno prossimo scenderà all'1 e altre cose che riguardano la vita dei cittadini e delle imprese italiane. Noi però, signor Presidente, riteniamo totalmente insufficiente la documentazione di accompagnamento all'emendamento del Governo che è stata trasmessa al Senato della Repubblica. Non si può presentare un emendamento che vale 10 miliardi di euro senza chiarire qual è il quadro macroeconomico *(Applausi l'economia di questo Paese, che nel frattempo sta scivolando verso la recessione, anche grazie alla vostra politica economica. E allora non ci possiamo accontentare delle dichiarazioni del *premier* Conte e delle dirette Facebook dei due Vice *Premier*. Noi chiediamo ufficialmente - lo abbiamo già fatto in Commissione e lo facciamo anche in Aula - che venga trasmessa al Parlamento una relazione di variazione della Nota di aggiornamento, come previsto dalla legge n. 243 del 2012, come è stato fatto nell'ottobre del 2014 dal Governo Renzi e come dovrebbe essere normale in ogni Paese civile, che quando presenta una manovra completamente diversa da quella che avete festeggiato...

Noi chiediamo di avere i numeri che avete dato a Bruxelles e non avete trasmesso al

il reddito di cittadinanza. Abbiamo il diritto di sapere quali promesse non saranno mantenute. E ce lo dovete mettere nero su bianco! Senatore Misiani, la legge che prevedeva quello che lei sta chiedendo è stata modificata nell'anno 2016,

era in ambasce, in attesa delle comunicazioni via etere dalla Commissione europea, quindi in balia se vogliamo dell'Europa. E lo dice mi avvalgo di essere senza vincolo di mandato, quindi non so se il mio Gruppo condivide pienamente - uno che sostiene che forse le regole europee vanno ridiscusse che, essendo noi un Paese fondatore, abbiamo tutto il diritto di chiedere la ridiscussione delle regole europee *(Applausi dal

anche l'opposizione ha rispettato il dovere della riservatezza rispetto alla trattativa che il Governo italiano svolgeva con l'Unione europea. Credo però che in una repubblica parlamentare,

i colloqui); non noi dell'opposizione, non noi singoli senatori ma il Parlamento italiano ne aveva diritto. Ciò non è avvenuto. Siamo qui senza aver votato nulla, come è già stato detto precedentemente. Siamo qui, peraltro, a discutere una manovra già vecchia, superata dai fatti pur essendo stata cambiata più volte. Ci fa piacere che non ci sia la procedura di infrazione. Il rapporto debito-PIL, che è stato tanto sbandierato al 2,4, oggi è al 2,04. Si tratta di 7 miliardi di euro per il nostro *deficit*, 7 miliardi di euro in meno che sono rilevanti ed importanti. Abbiamo comunque 1,7 miliardi in più di margine rispetto al 2 per cento che era la somma tra il tendenziale e le clausole di salvaguardia precedenti

Questo è il risultato di una manovra che è peggiorata. Praticamente siamo passati dalla dalla manovra di cambiamento al cambiamento della manovra, anche se la frase non è mia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. La prima domanda che ci siamo posti, quindi, è se le due misure ritenute prioritarie che questa maggioranza ha mantenuto siano più importanti di altri interventi volti alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro, perché l'indicazione che è sempre venuta era favorevole alla crescita, ad una manovra espansiva. Poi ci siamo posti l'interrogativo se una volta fatti quadrare i conti con l'Europa solo per il 2019 il problema sia risolto anche per i prossimi anni. La risposta è no. Chi farà la manovra del 2020 e del 2021 in questo quadro? Siamo infatti in presenza di una semplice posticipazione dei problemi, dei debiti e naturalmente degli indicatori. Siamo con le due misure principali totalmente a debito, spese di parte corrente continuative non *una tantum*, quindi ci troveremo dal 2020 ad avere continuativamente questo tipo di spesa. Il dato politico più sostanziale - permettetemelo - è forse la sconfitta del balcone, di quella parte della maggioranza che si è affacciata al balcone, dei 5 Stelle e delle loro promesse elettorali da 17 miliardi

Questa potrebbe essere la manovra di un vero Governo che ha a cuore le sorti della Nazione. Forse - e concludo dobbiamo ringraziare la Banca centrale europea, che nonostante la riduzione graduale del piano di acquisti ha confermato il riacquisto dei titoli in scadenza attualmente già in portafoglio. una manovra recessiva che plasma l'idea della decrescita felice, mentre questo Paese ha bisogno di creare ulteriori condizioni di crescita del lavoro e ulteriori opportunità

l'Europa, che ci sarà un *deficit* inferiore a quello preannunciato e che, comunque, i provvedimenti che la maggioranza riteneva importanti, come il reddito di cittadinanza, saranno mantenuti.

Detto questo ci preoccupiamo perché dalle parole che il Presidente del Consiglio ha detto ieri abbiamo fondamentalmente capito una cosa: il Governo italiano è andato a Bruxelles e ha chiesto la possibilità di fare la sua manovra elettorale in vista della prossima campagna per le europee in cambio in cambio di un'ipoteca nei prossimi anni sul futuro dei nostri cittadini. Quello che succederà, come qualcuno ha già detto, nel 2020-2021 non è ancora chiaro.

ad oggi, non ci consente di capire ancora quali siano effettivamente i dati su cui discutere.

in esso elementi di sviluppo, possibilità di aumentare i posti di lavoro. O meglio, i posti di lavoro effettivamente li avete creati nella manovra. Li avete creati quando,

sono *una tantum*, quindi voi cosa volete fare con questo provvedimento? Volete sostituire delle spese *una tantum* con una spesa strutturale che sarà sempre

come dite, dei posti di lavoro. Come? Con il reddito di cittadinanza? Gli unici posti di lavoro che creerete saranno molto probabilmente i 4.000 destinati ad ampliare i centri dell'impiego. Quelli sì, sono posti di lavoro certi. Però ancora non avete capito una cosa: il problema dei centri per l'impiego non è la quantità delle persone

voluto abolire di fatto, rendendo la situazione istituzionale pazzesca - avrebbe capito che i centri per l'impiego non funzionano perché non c'è una selezione vera del tipo di lavoratori che servono al territorio. Molte volte all'interno dei centri per l'impiego, e di quelle che erano prima le Province, venivano fatti i corsi di formazione che non avevano neanche un'attinenza minima con il lavoro che

i lavori da fare all'interno dei porti e la manutenzione straordinaria. Si potrebbe continuare ancora, ma voglio andare nello specifico di una materia che mi interessa particolarmente, quella dell'agricoltura. In questa finanziaria - almeno stando a quello che ci è dato sapere - per l'agricoltura, che rappresenta uno degli *asset* fondamentali delle nostre esportazioni, del *made in Italy*, dell'agroalimentare, avete investito zero; avete investito lo zero virgola Avete investito circa un milione l'anno per il problema della *xylella fastidiosa* in Puglia. A fronte di stime da parte della Coldiretti, della Confagricoltura e delle

Avete detto che investite 10 milioni di euro per la forestazione? Ma vi rendete conto? 10 milioni su più di 11 milioni di ettari di boschi che abbiamo nel nostro Paese? Non è neanche un euro a ettaro. E se anche dovesse essere suddiviso per Comuni, non per ettaro, considerato che abbiamo 3.500 Comuni montani nel nostro Paese, non viene neanche una media di 3.000 euro a Comune. Quindi con quali soldi volete aiutare l'agricoltura italiana? L'ultima cosa. La vostra operazione di bandiera in agricoltura era quella di regalare un ettaro di terra a chi avesse il terzo o il quarto figlio? Ma di cosa state parlando?

questa, per quello che c'è stato dato di vedere fino ad oggi, è una manovra che non fa crescere l'occupazione, che non crea sviluppo, ma crea solo assistenzialismo. Per quanto ci riguarda, avremmo voluto una manovra più italiana, più patriottica, meno europea. Ma mi sembra che la vostra rivoluzione, che avete annunciato dai balconi, si stia nascondendo nelle cantine della politica.

il disagio di chi, per cultura, per tradizione, per pratica, ha fatto del rispetto delle istituzioni il punto cardine della sua attività politica. Prendo la parola con disagio, perché a me pare che oggi compiate, in questi giorni già così cupi, un ulteriore grave attacco, il più grave nella storia della nostra Repubblica,

Vedete, che il Parlamento sia umiliato, esautorato, ridotto all'irrilevanza, anzi - consentitemi non è un trofeo di cui andare orgogliosi, non è un *vulnus* all'opposizione, ma è una ferita grave a tutti,

Alla Camera avete preteso, con la fiducia, la votazione su una manovra farlocca che tutti sapevamo non esistere (lo leggevano ogni mattina). Qui pretendete, allo stesso modo, una votazione con la fiducia su un oggetto misterioso che nessuno ha avuto la possibilità, oltre che il dovere, di esaminare. Il presidente Conte ieri ci ha dato alcune cifre, ma mi pare che più che altro da molti vengano dati i numeri e dare i numeri non è sinonimo di partire dalle cifre: è dare i numeri.

in termini politici, di credibilità del nostro Paese e in termini economici per gli italiani, le italiane e le famiglie di questo Paese. I costi politici non li recupererà più nessuno e il tutto in questi mesi è stato accompagnato da esternazioni giornaliere dei due vice, Salvini in particolare, irrispettose, da bullo di periferia, volgari quando non direttamente insultanti verso chiunque. Se un magistrato osa dire che a indagini aperte sarebbe bene non twittare, gli si risponde che è stanco e che vada in pensione. Se un alto funzionario prova a dire che i numeri sono una cosa e le cifre macroeconomiche sono altro, gli si risponde in modo sprezzante che si faccia eleggere e poi parli perché «noi siamo eletti da 60 milioni italiani», e non è vero, e FI-BP)*. E comunque, con 60 meno uno e sono contenta, per lo meno, di capire quali sono le nostre differenze di fondo sulla gestione politica e liberale di un Paese come si deve. E vogliamo continuare su «Tanti nemici tanto onore» oppure «Tireremo dritto», oppure «Cacceremo 500.000 clandestini», con cui ci avete rintronati per mesi di campagna elettorale? Salvo che tra una birreria e una bocciofila, a un certo punto il Ministro dell'interno ha avuto persino il tempo di passare al Ministero e qualcuno gli ha suggerito che non era possibile - glielo dicevamo da mesi - e ha dovuto ammettere che in effetti ci vorrebbero ottant'anni.

una penosa e silenziosa retromarcia, per nostra fortuna e per fortuna dell'intero Paese. Paese. A chiunque abbia potuto evitare che il vagone Italia precipitasse nel burrone, va il nostro apprezzamento e quello dell'intero Paese. Eravamo vicini al burrone e io, che non apprezzo per cultura il «Tanto peggio tanto meglio», devo anche dire che non precipitare nel burrone è un valore per tutti e anche per questo Paese. Nel merito, molto è stato detto. Colleghi, è veramente bizzarro, per non dire di peggio,

È una bella scoppola! Capisco le assenze di Salvini e di Di Maio ieri: uno impegnato in famiglia e poi in birreria, e l'altro sicuramente in grandi attività. Ma, dopo tutte le limature per ben 10 miliardi - alla faccia delle limature - questa rimane una manovra spendacciona in spese correnti, una manovra elettorale che non affronta affatto i problemi reali di questo Paese. Un doppio sfregio: uno sfregio istituzionale e uno sfregio per il rilancio del Paese. del Paese. Per onorare quello che rimane di questa democrazia parlamentare, sono seriamente tentata di non partecipare al voto;

attaccamento ho alla democrazia aperta, alla democrazia liberale; quella democrazia che mi sembra il modo meno peggiore di governare un Paese.

ma quello che resta sono esattamente gli equilibri di potere tra i vari ruoli. Qui non c'è neanche più la differenza tra l'esecutivo e il giudiziario

*(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è difficile rimanere insensibili all'intervento di chi mi ha preceduto, che dimostra tutto l'attaccamento alle istituzioni, al ruolo, alle funzioni alle quali siamo votati e che dobbiamo rispettare e onorare anche in quest'Aula. nella mia non breve esperienza parlamentare, signor Presidente, non mi era mai capitato che si arrivasse a discutere di un manovra finanziaria senza che la Commissione

quando sarà presentato il maxiemendamento, ci darete due ore per i subemendamenti, quando voi, in tre mesi, ancora non siete stati capaci di varare una manovra finanziaria.

Vede, signor Presidente, abbiamo visto la differenza qualche minuto fa: pur non essendo responsabilità dell'opposizione il ritardo con il quale arriveremo a votare la manovra finanziaria, pur non conoscendo ancora nei dettagli e precisamente quali saranno le poste cambiate, quali saranno gli interventi aggiuntivi e quali verranno sottratti, abbiamo proposto, non in maniera provocatoria,

quando da quel balcone, battendo i pugni sul petto, si diceva: «Abbiamo varato la manovra del popolo, con il 2,4 per cento di *deficit*, in cui ci sono tutte le risorse e tutte le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale. Noi non andremo in Europa con il cappello in mano!». No, voi siete andati in ginocchio e avete fatto pagare un prezzo altissimo al Paese!

Come già successo ad altri autorevoli esponenti politici prima di voi, arriva sempre il giorno del giudizio e non quello universale, ma quello popolare. Forse riuscirete anche a raggiungere il vostro obiettivo alle elezioni europee,

Per varare questa manovra e per avere l'autorizzazione da parte dell'Europa, che non è un atto di fede, ma è un'autorizzazione subordinata, a gennaio vi chiederanno di vedere i compiti che avete fatto

voi sapete che non governerete in quel tempo. Voi volete soltanto rubare un consenso alle elezioni europee e andare a casa, perché andrete a casa, o di vostra volontà o mandati dal popolo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Saranno altri ad assumere la responsabilità di tirare dalle secche il Paese che voi avete portato in queste condizioni. Allora mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che nella mia terra, nella mia Regione e in tutto il Sud, hanno fatto incetta di voti, hanno preso tutti i collegi uninominali promettendo scintille a favore del Mezzogiorno. Voi avete una grande responsabilità e di questa responsabilità un giorno sarete chiamati a rendere conto.

di rappresentare e difendere il Mezzogiorno. Noi saremmo stati dalla vostra parte, perché saremmo stati dalla parte dei più deboli e dalla parte del Mezzogiorno. E voi che cosa avete fatto? Dov'è finito il credito d'imposta? Come pensate che si possa sviluppare l'economia e possa aumentare l'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia? Avete tagliato 800 milioni per i fondi di solidarietà sociale; avete tolto tutti gli ammortamenti. Pensate che al Mezzogiorno basti un rivisto reddito di cittadinanza o qualche elemosina di questo tipo? Non conoscete i meridionali! Noi potremo essere anche poveri, ma abbiamo un

al reddito di cittadinanza, a voi che andate sui giornali, sulle piazze e sui *social network* a dire che tutte le promesse sono mantenute, ricordo che eravate partiti da 9 miliardi, sono rimasti 7; togliamone uno per i centri di occupazione e ne sono rimasti 6. La platea di poveri assoluti del nostro Paese è formata da 5 milioni di italiani; dividendo i 6 miliardi per i 5 milioni di poveri viene forse qualcosa in meno di quei famosi 80 euro che sono stati drammatici per qualchedun altro e che segneranno lo stesso destino anche per voi.

Signor Presidente, signori del Governo, vogliamo denunciare il vostro comportamento di queste settimane di continua offesa del Parlamento, quindi del Paese,

alla Camera, una manovra completamente infondata e in larga parte falsa. Non avete avuto remora a prendere in giro il Senato della Repubblica per giorni e giorni, impedendo che ci fosse anche un solo voto di merito nella Commissione bilancio. Non avete remore, ancora in queste ore, a farci discutere quando ancora state manomettendo una manovra che è come un gioco delle tre carte. Noi, signori del Governo, vogliamo denunciare queste continue vostre sceneggiate, questa continua vostra irresponsabilità che sta costando un prezzo altissimo per tutti gli italiani, soprattutto per chi è più debole. Ma a voi di questo, a quanto pare, non interessa nulla. A voi non interessa la vita reale e quotidiana. Voi vivete sui *social*, negli studi televisivi. La vostra è una continua finzione. Sono passati tre mesi da quella pantomima inquietante del balcone di Palazzo Chigi, quando, offendendo ed umiliando milioni di persone che ogni giorno lottano onestamente tra mille difficoltà, il vice presidente Di Maio,

uno *spread* fuori controllo. E non è teoria, ma pratica concretissima. Significa oltre un miliardo e mezzo, che stiamo già pagando, in aumento dei mutui per le famiglie, prestiti per le imprese, in aumento delle bollette di luce, acqua e gas*.* È vita reale, signori del Governo. Ma a voi non interessa. In questi mesi di bullismo, di sbruffonerie sbruffonerie è crollata la fiducia, sono scappati gli investitori, sono diminuiti i consumi, sono calate le nostre esportazioni, le quote di mercato del nostro *made in Italy*. Il nostro Paese è più debole e più difficile è la prospettiva per milioni di lavoratori, di artigiani, di imprenditori e per la prima volta dal 2014, dopo quattordici trimestri consecutivi positivi il nostro prodotto interno lordo scende. Voi ci state precipitando nella recessione! E a pagarla non saranno i forti, quelli con le spalle coperte. Voi la farete pagare ai più deboli. Lo sappiamo. Lo avete scritto voi questa notte, perché i dieci miliardi di tagli che costa la vostra ridicola ritirata dall'Europa li trovate aumentando l'IVA, cioè la tassa che tutti gli italiani pagano quando fanno la spesa per mangiare; li trovate tagliando le pensioni di 1.500 euro lordi, signori del Governo, colpendo il ceto medio e lasciando indisturbati i forti e gli speculatori. risorse agli enti locali, ai Comuni, alle città, alle periferie. La vostra è una manovra tutta imperniata su un assistenzialismo farlocco, ingannevole, che non salva, che non protegge, che non emancipa, ma che invece ghettizza, esclude. Il vostro, infatti, non è un reddito di cittadinanza, ma una mancia di povertà,

da difendere e da creare: ma qui non c'è nulla; è investire nell'istruzione: ma qui non c'è nulla. Non c'è nessuna idea di futuro in questa manovra, che imponete con l'ennesimo voto di fiducia, strozzando le regole e impedendoci anche di parlare, mortificando questo Parlamento. Diritto allo studio, ricerca, università, che sono il nostro futuro e che determineranno il posto dell'Italia nel mondo: voi, da questa legge di bilancio, che è la carta d'identità del Paese, li fate scomparire.

che sono briciole offensive. Il vostro è l'incremento più basso dal 2012. Voi stoppate una crescita continua che, negli ultimi anni, ha portato quasi a raddoppiare il fondo per le borse di studio e per il diritto allo studio. Voi cancellate

per la prima volta dai tempi di Tremonti (siete gli epigoni di Tremonti!), voi per la prima volta causerete una diminuzione dei finanziamenti al sistema dell'università e del diritto allo studio. Togliete lo avete fatto questa notte - 100 milioni alla ricerca; togliete 300 milioni al credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione; togliete l'indicizzazione del 3 per cento a quel fabbisogno universitario che voi, invece, volete legare alle stime del PIL. Ma lo sapete che sono molto più basse, molto inferiori e questo causerà un definanziamento strutturale per i decenni a venire! Questa è una norma devastante anche sul piano simbolico, perché significa retrocedere l'università dalle priorità del Paese.

uno schiaffo in faccia, un colpo alla schiena a tantissimi giovani, che spezza vite, carriere e umilia anni e anni di lavoro e rigetta nel precariato. Impedisce anche di maturare trattamenti previdenziali; vanifica quello sblocco del *turnover* conquistato faticosamente in questi anni. Dico: fermatevi; non mortificate una generazione di studiosi. Voi avete bocciato tutti i nostri emendamenti

fattibili per affrontare i grandi mali della nostra università, che sono il precariato nella ricerca, la scarsità… PRESIDENTE. Senatore Verducci, la ringrazio. Vorrei che rispettassimo i tempi visto che finiamo a mezzanotte. Le ho dato un minuto in più.

*(PD)*. Sono accalorato per questi mali: la precarietà nella ricerca, la scarsità di immatricolati e laureati, le disparità territoriali stati abbastanza contrastati in questi anni, ma che risalgono agli anni di Tremonti e Gelmini. Del resto, voi, signori del Governo, i protagonisti di quella stagione buia, come Valditara, li avete messi oggi di nuovo a comandare l'università italiana. Allora di che parliamo? Il vostro è un passo indietro oltraggioso; avete tradito aspettative, fatto carta straccia di promesse. Di questo dovreste vergognarvi; anzi, di questo già vi vergognate, visto che il vice ministro Fioramonti pochi giorni fa alla Sapienza ha detto testuale:

un vero atto di accusa contro il vostro Governo. In questi giorni di mobilitazione nelle scuole e nelle università hanno detto: non vogliamo condoni che significano criminalità; non vogliamo sussistenza che svilisce la nostra dignità; vogliamo solidarietà; vogliamo scuola pubblica; vogliamo lavoro. Hanno ragione e se vinceranno - e vinceranno - avrà vinto l'Italia. Noi faremo valere in questa Aula e nel Paese la nostra voce, a fianco di quella voce, per questo nostro Paese, che non permetteremo a nessuno di mortificare, come state facendo.

adusi a trattare Governi eletti dal popolo sovrano come i loro più fedeli camerieri, approveremo la legge di bilancio, arrivata in Senato dopo un percorso accidentato, una corsa a ostacoli della cleptocrazia europea

con la rivoluzione mite delle matite. I mercati - disse quel signore - insegneranno agli italiani a votare. Il 23 maggio un lancio dell'agenzia Reuters

da ministro delle finanze francese, tra il 2012 e il 2014 aveva criticato la politica di austerità e il rigore imposti dall'Europa alla Francia. Altri periodici anatemi venivano lanciati contro il Governo da Dombrovskis, dal ministro delle finanze francese Le Maire, rammaricato che l'Italia non avesse accettato i *Diktat* della Commissione europea, forse per soddisfare gli antichi appetiti sulle aziende pubbliche italiane, come la Germania aveva fatto in Grecia. In ultimo, il presidente Juncker, alla domanda sul perché in diverse occasioni avesse chiuso un occhio sulle infrazioni francesi, ha ammesso di averlo fatto perché è la Francia,

Eppure lì c'è stata la rivolta e voi dovete ringraziare il MoVimento 5 Stelle e la Lega, perché qui non sono arrivati i gilet gialli *(Applausi dai Gruppi

e Moscovici, (conflitto d'interesse?) ha detto che lo sforamento è possibile in quanto limitato. Agli smemorati che si agitano contro il Governo MoVimento 5 Stelle - Lega, invece di essere uniti sulla tutela dei diritti e degli interessi dell'Italia, voglio ricordare che tra i 28 Paesi dell'Unione europea, poco più di uno su due nel 2016 non ha rispettato le disposizioni previste dai principali criteri.

e in tale disastroso strabismo di commissari europei che odiano palesemente questo Paese, odiano l'Italia ed il suo legittimo Governo, la manovra del popolo che ci accingiamo a votare contiene reddito e pensione di cittadinanza, pensionamenti anticipati, quota 100 per correggere la sciagurata legge Fornero,

Io, signor Presidente, mi accingo a chiudere, perché un'Unione europea che ricatta i popoli che non votano secondo i suoi *desiderata* e fa dipendere la propria sopravvivenza da uno 0,4 in più o in meno, che si affanna a far valere una sorta di sovranità economica favorevole per gli Stati amici, come la Francia, contraria per l'Italia, loro nemica, sol perché il popolo sovrano non ha votato secondo i desideri della cleptocrazia europea, quest'Europa non può avere futuro. E l'ansia dello *spread*, la manipolazione mediatica delle coscienze dei professionisti dell'angoscia sul pericolo grave dei sudati risparmi degli italiani, da chi arriva? Dagli Dagli Attila dei risparmiatori, da quelli che hanno truffato 500.000 famiglie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vi ricordate il Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza? Ossessivamente ripetute decine di volte al giorno. Ebbene, alle parole in libertà di chi, tra le più alte cariche, avrebbe il dovere di difendere il bene comune e l'interesse generale, invece delle risibili magliette sbiadite di partiti *desaparecidos*, noi del MoVimento 5 Stelle contrapponiamo i valori della Costituzione, che abbiamo difeso il 4 dicembre contro il *referendum* J.P. Morgan. La sovranità appartiene al popolo, non allo *spread* e ai banchieri, che vorrebbero renderci loro moderni schiavi. Chiudo, signor Presidente. Noi, che governiamo da soli sei mesi, cercheremo in cinque anni di ripianare e riparare i gravissimi disastri che avete procurato in vent'anni. *(Applausi dal

Poiché è prevista la chiusura alle ore 24, spero mi aiuterete nel rispetto dei tempi,

Presidente, Governo, colleghi senatori, intervengo su un disegno di legge di bilancio che ancora non c'è, dando atto oggi al Governo e a questa maggioranza di aver mantenuto un impegno. Avevate promesso di scrivere la storia e ci siete riusciti: mai nella storia repubblicana, infatti, una manovra finanziaria era arrivata con tanto ritardo alla conoscenza del Parlamento. Mai era accaduto

Questa sarà la vostra storia e per questo sarete anche ricordati in futuro. A un passo dall'esercizio provvisorio del 31 dicembre, ancora oggi non conosciamo il contenuto della proposta di legge, la più importante per il Paese, l'atto politico per eccellenza

Perché le proposte che avete fatto fino a oggi erano poco serie e non erano assolutamente fattibili, per quanto riguarda sia la spesa, sia le misure che avete presentato all'Italia e all'Europa. Quindi una proposta assolutamente non credibile, ma zeppa di misure irrealizzabili; e infatti è stata stroncata. Non voglio soffermarmi sulle vicissitudini di questa manovra finanziaria, che è stata sicuramente tormentata. Siamo partiti dalla sfida di sforare il 3 per cento, per poi passare a sfiorare il 3

Nel frattempo, però, i nostri cittadini, gli italiani, i portafogli, le nostre famiglie e le imprese hanno perso 250 miliardi di capitalizzazione, di investimenti delle nostre famiglie che avete bruciato

dello sbandierato sovranismo, l'esito è stato fallimentare. Per giungere a una resa incondizionata con l'Europa il passo non è stato breve e nemmeno indolore. Abbiamo avuto mesi di *spread* a livelli altissimi e oggi le conseguenze le pagheranno le nostre famiglie perché dalle prossime settimane troveranno i tassi per mutui e prestiti più alti presso gli istituti di credito. Tutto prevedibile, ma il Governo ha voluto comunque sfidare l'Europa non soltanto l'Europa ma soprattutto il buon senso. La prova che la strada intrapresa fosse impraticabile e dannosa per gli italiani è nel commento che anche voi del Governo fate oggi, perché ritenete che la manovra sia stata persino migliorata, perché è diventata più prudente e perché alla fine ha vinto il dialogo: sono dichiarazioni del Governo. Quindi a che gioco abbiamo giocato fino ad oggi? Abbiamo giocato mettendo le mani nelle tasche dei cittadini quando, invece, con arroganza, ci siamo isolati dal contesto europeo. Si sono sparate cifre a caso e si sono proposti anche indebitamenti colossali che avrebbero pesato per decenni soprattutto sulle giovani generazioni, per poi dover alla fine ringraziare l'Europa dopo averla denigrata.

La manovra, quindi, è stata riportata sui binari della sostenibilità finanziaria e allora, a settembre, sul balcone di Palazzo Chigi, che cosa abbiamo festeggiato? Quale vittoria abbiamo festeggiato allora? Di sicuro avete festeggiato la vostra superbia che, come sempre nella vita, parte a cavallo e torna a piedi. vi invito a ritornare su quel palazzo, sul quel balcone soprattutto, e chiedere scusa agli italiani per i danni che avete arrecato in queste settimane, in questi mesi di trattative. Avete fatto una magra figura, la figura degli adolescenti, di quegli adolescenti che oggi sono contenti di aver disatteso, di aver trasgredito qualche regola. Ma voi non siete adolescenti perché voi oggi rappresentate il Paese, perché voi oggi siete al Governo e avete una responsabilità importante e - ahimè - invece, in questa trattativa, oggi, a rimetterci sono stati proprio gli italiani ma soprattutto quel popolo con cui tanto riempite la vostra propaganda. quali sono stati e quali sono i brillanti risultati di questa manovra che, come dicevo, non c'è ancora ma leggiamo dai giornali? Alla fine, siamo scesi

Quindi di quale manovra espansiva parlate se alla fine, dall'1 per cento, passeremo nel 2019 all'1 per cento? Queste sono barzellette e anche se le raccontate come barzellette, queste cose non fanno assolutamente ridere. Non c'è nessuna manovra espansiva e gli italiani lo devono sapere perché i numeri sono questi. Siamo ad un passo dal 31 dicembre, quindi dal rischio dell'esercizio provvisorio, però, nello specifico, noi oggi abbiamo 4 miliardi in meno di investimenti, 2 miliardi di fondi congelati a garanzia del *deficit* strutturale, un rapporto

lo stop alle indicizzazioni in aumento delle pensioni a 1.500 euro. Questa è una vergogna e la pagherete davanti ai cittadini. *(Applausi dal

mettete il genio militare a tappare le buche di Roma. E proprio di Roma dobbiamo parlare, come ha fatto in modo documentato proprio ieri l'ISPRA, che ha presentato la sua indagine 2018 sulla qualità dell'ambiente urbano, fornendo dati e cifre sul dissesto idrogeologico, sull'erosione, sulle frane e sulle alluvioni. Il rapporto denuncia a Roma un *boom* di buche; 136 voragini negli ultimi dieci mesi dell'anno in corso. Premesso che a Roma la vera emergenza è il suo sindaco,

un biennio, che coincide esattamente con la fine del mandato dell'amministrazione capitolina. Insomma, nella manovra finanziaria abbiamo fatto passare una misura salva Raggi. Ma non è solo questo che

e rattoppare come in questo caso. Ha ragione allora Giorgia Meloni quando con una battuta, forse anche per sdrammatizzare questa manovra drammatica, dice che dalle truppe d'assalto siamo passati alle truppe d'asfalto: purtroppo è così.

parla indistintamente e genericamente di un taglio di un miliardo di spese inutili che andranno ai centri per l'impiego. Quali siano i tagli non è ancora chiaro, per ora sappiamo con certezza - e lo voglio dire con molta chiarezza - che i tagli vanno alla ricerca, allo sviluppo, alla difesa e alla sicurezza:

Voglio ricordare agli estensori della manovra che l'esercito nasce per difendere le Istituzioni, i cittadini, i confini e la pace istituzionale non nasce per coprire le buche di chi non ha saputo gestire. L'esercito italiano è una delle quattro Forze armate: non vi vengono i brividi quando scrivete queste cose? Non pensate all'esercito regio nato nel 1861 Non pensate all'esercito italiano nato con la Repubblica italiana nel 1946? Non pensate all'esercito italiano, una delle quattro Forze armate impegnate nell'Alleanza atlantica e nelle missioni di *peacekeeping*, di stabilizzazione, di deterrenza dei rischi rischi globali? A che pensate quando dite le parole esercito e genio militare? Non pensate alla realtà. Non mi stupirei se un giorno mandaste la fanteria a raccogliere i pomodori! Nella migliore delle ipotesi, nella vostra manovra c'è un'ottica perversa che vuole trasformare l'esercito in una specie di Protezione civile allargata: l'esercito è nato con altri compiti, ha un'altra storia e deve avere un altro impiego. Io non voglio vedere un militare con la sua mimetica, definita tuta da combattimento, a tappare le buche di chi non ha saputo lavorare. Questo succede perché gli estensori della manovra non hanno il senso dello Stato e delle Istituzioni. Quando parlate di manovra del popolo mi ricordate i Giacobini, quelli della terza fase però, quelli dei Robespierre per capirci: andate andate a studiare le distinzioni di Michelet sulla terza fase di giacobinismo. Non amate lo Stato, non rispettate le Istituzioni e questa manovra è una manfrina elettorale. Avete prima mostrato i muscoli, avete fatto i gradassi e poi avete fatto marcia indietro su tutto e sapete - perché lo sapete - che avete messo insieme non una sintesi, ma una somma di misure e di mancette elettorali prive di una visione di insieme, di di un progetto, di un orizzonte, di un piano di sviluppo. Ebbene, con questa manovra non si va lontano.

Signor Presidente, colleghi senatori, ringrazio i colleghi di Commissione per il lavoro svolto, i rappresentanti del Governo per il confronto costruttivo e i colleghi

che oltre a contenere misure economiche per lo sviluppo del nostro Paese, contiene provvedimenti significativi per i nostri Comuni. Da sindaco di un piccolo paese della bassa veronese, il Comune di Concamarise, confido nel Governo, che potrà mettere in atto alcune richieste avanzate dai sindaci, presentate attraverso gli emendamenti. Alla mia anticipazione, nei giorni scorsi, della possibilità di queste misure ai sindaci del mio territorio,

ma anche da molti altri sindaci di estrazioni politiche diverse dalla mia, anche da sindaci rappresentanti per la quasi totalità dei gruppi politici presenti in questo Parlamento, anche da sindaci del Partito Democratico

per quei sindaci dei Comuni che vivono per la gente e con la gente. Sindaci che respirano i sentimenti delle comunità che amministrano, che siano sentimenti positivi o negativi. Di seguito elencherò le principali misure che potrebbero andare in vigore nel 2019 e che riguardano i Comuni italiani uso il condizionale perché il Parlamento nelle prossime ore sarà chiamato a votare tali misure: modifiche significative alle regole di finanza pubblica relative agli equilibri di bilancio in riferimento all'utilizzo degli avanzi di amministrazione a seguito delle recenti pronunce della Corte costituzionale; possibilità di richiedere anticipazioni di tesoreria per accelerare il pagamento dei debiti commerciali; incremento delle risorse per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici pari a 25 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022; contributi per 400 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; semplificazione degli adempimenti contabili. le società a partecipazione pubblica che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente non verranno messe in liquidazione; revisione del codice degli appalti senza gara per gli importi inferiori a 200.000 euro. Con queste misure, tra l'altro, daremo la possibilità di cantierare immediatamente i lavori pubblici facendo lavorare le aziende del territorio e

per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quei Comuni che spesso vivono la difficoltà delle chiusure degli uffici postali, che con questa misura possono dar vita agli uffici postali nei propri Comuni. Concludo aggiungendo che siamo consapevoli che da parte di tutti si vorrebbe fare di più. Ma, come ho più volte detto in questi miei nove anni da sindaco, non abbiamo la bacchetta magica. Stiamo operando con umiltà verso idee concrete.

Non siamo quelli del nuovo miracolo italiano, non siamo quelli che hanno promesso agli italiani che, entrando in Europa, si sarebbe lavorato cinque giorni alla settimana. Non usiamo lo stile delle promesse del "bomba" con il motto «l'Italia cambia verso», che contrapponeva il futuro alla conservazione.

dovendo scendere nelle strade, insieme ai nostri compaesani, a manifestare, manifestando contro la vostra volontà di svilire i nostri territori. Noi siamo qui per lavorare a testa bassa...

Signor Presidente, la legge di bilancio che la maggioranza si accinge a ratificare - con un dibattito parlamentare completamente annichilito, costellato di veri e propri inediti, poggiato su una discussione finta, impapocchiata tra improvvisazione e cose non dette - segna la definitiva consegna delle sorti del nostro Paese alla penna dei burocrati di Bruxelles. È una legge di bilancio che viene sottoscritta da sovranisti senza sovranità e che, per paradosso, non ci sottrae totalmente al rischio di procedura di infrazione, e dunque ad un periodo di nuova e più dura austerità. La manovra scritta a Bruxelles, però, pone fine al teatrino - e questo forse è l'unico fatto positivo - delle stime di crescita giudicate inattendibili da tutti gli istituti internazionali e impone una riduzione del *deficit* di almeno 11 miliardi, pari ad una correzione dello 0,6 per cento del PIL. Mi chiedo allora: perché avete festeggiato sull'ormai famoso balcone di Palazzo Chigi l'intesa al 2,4 *deficit*-PIL, se oggi quell'intesa - qui nel testo in votazione - non c'è più? Perché avete esultato per l'avvenuta abolizione della povertà, quando oggi, con questo testo in discussione, lo scenario descritto ci consegna ad una prospettiva di decrescita e quindi ad un inevitabile aumento della povertà relativa? Con tipico tratto da spacconi, imbevuti di celodurismo immaginavate di ricevere la letterina di Babbo Natale.

con tipico tratto da spacconi, imbevuti di celodurismo immaginavate di ricevere la letterina di Babbo Natale e, invece, consegnate per vostra mano al Paese una lettera con cui la Commissione europea vi costringe al ritorno ad un *deficit* di 1,8, alla situazione di settembre, con un taglio di 0,6 punti che oggi però disvela, davanti a un calo del PIL, un aumento del peso di quello stesso *deficit* sul Paese. Tornate dunque al più ragionevole rapporto del 2 per cento, ma in due (o forse tre?) mesi vissuti a colpi di *post*, *tweet* e foto con i gattini, avete fatto bruciare qualcosa come 300 o 400 miliardi di risparmi e di ricchezza agli italiani, avete fatto pagare un conto di almeno 1,5 miliardi di euro di maggiori oneri per la gestione del debito per via di uno*spread* che era arrivato alle stelle e che nemmeno la vostra approvazione riuscirà ad addomesticare. Ma questo, purtroppo, non è il conto finale della vostra incompetenza. Purtroppo non è tutto. La riscrittura fatta a Bruxelles, conseguenza di questa vostra irresponsabilità, ci consegna una manovra recessiva in cui non vi sono misure per la crescita, spariscono gli investimenti, vengono penalizzate le imprese, mortificato il Sud con pesanti tagli ai cofinanziamenti ai fondi regionali, bloccato il *turnover* nella pubblica amministrazione, e finalmente smascherata la propaganda di reddito di cittadinanza e quota 100, dei quali resta qualcosa più del titolo e l'assoluta incertezza dei tempi di attivazione. Ecco, quindi, spiegati i tagli per circa 11 miliardi di euro nel 2019: tagli, non risorse aggiuntive. Tra queste, urla vendetta la indicata riduzione di almeno 700 milioni di fondi per le Regioni, già stanziati per cofinanziare fondi strutturali dell'Unione europea, destinati alla realizzazione di interventi di mitigazione dei rischi ambientali e idrogeologici. Altro che salvaguardia del territorio! Urla vendetta il taglio di 800 milioni di euro dalla riprogrammazione della cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione altro che Ministro per il Sud! Urla vendetta il taglio di 850 milioni di euro alla rimodulazione dei fondi di cofinanziamento nazionale. Un martirio vero e proprio che vale almeno 2,5 miliardi. Ma non Ma non basta ancora. Anziché concentrare risorse per accompagnare i chiari segnali di crescita registrati sino all'avvio di questo Governo, con vero e proprio masochismo si escogita un taglio di ulteriori 410 milioni che va a colpire direttamente le agevolazioni alle imprese, attraverso i quali limate il credito d'imposta IRAP e azzerate totalmente il credito di imposta per per l'acquisto di beni strumentali nuovi; tagliate i fondi delle agevolazioni Ires e, poi, giusto per farsi male fino in fondo, vi producete anche in un taglio che riduce lo stanziamento di risorse per il capitale immateriale. State operando per la desertificazione economica del tessuto produttivo del nostro Paese, con una manovra che si legge al contrario: una vergogna. Ma non basta. Avete dovuto accettare anche l'inserimento di una clausola di salvaguardia di almeno due miliardi di euro, a garanzia del rispetto dei conti nel 2019: una vera e propria fideiussione - questa volta sì, innovativa - nella prassi dei rapporti tra Unione europea e Stati membri, a garanzia di un pagatore di cui ormai non si fida più nessuno. Questo è il risultato delle scarpe dei vostri eurodeputati che schiacciano i documenti della Commissione europea, questo è il risultato dei vostri «tireremo dritto» e «me ne frego», il risultato della vostra spocchiosa arroganza, con cui vestite una campagna elettorale perenne, che dura troppo, troppo a lungo, insopportabile e irresponsabile. Ripeto: la manovra che siete costretti a votare è strumento di politica economica recessiva, orfana di qualsiasi misura volta alla crescita. Altro che «manteniamo tutti gli impegni» o «avevamo solo esagerato nelle previsioni di spesa»: siete incoscienti consapevoli. C'è un ulteriore fatto che preoccupa fortemente: l'assenza di spazi di flessibilità sull'intero triennio 2019-2021, perché il Governo li ha già ipotecati tutti. Sì, perché il Governo ha fatto saltare lo schema per cui le clausole IVA potevano essere fatte slittare di anno in anno, usando per larga parte la flessibilità. Sino a oggi si poteva fare, da oggi non più. Nel 2020 o l'IVA aumenta di 3,5 punti percentuali oppure la si dovrà coprire con altre tasse o altri tagli particolarmente gravi dal punto di vista della sostenibilità politica e ancor di più economico e sociale. La principale differenza rispetto alle altre manovre - lo dico anche a qualche mio collega di Commissione che si qualifica economista - è che questa volta si è scelto di utilizzare per intero la flessibilità e per tutto il triennio; di sprecarla, di lasciarci senza protezione. In passato la flessibilità si otteneva sull'anno successivo e si mantenevano così obiettivi importanti di riduzione del *deficit* strutturale per gli anni successivi. Questa volta no: è già previsto che la discesa del *deficit* strutturale sia minima sul 2020 e sul 2021, quindi l'anno prossimo si avranno clausole IVA per almeno 23 miliardi di euro e per almeno 29 miliardi di euro nel 2020, con una flessibilità che, nel migliore dei casi, non potrà superare lo 0,2 per cento. La cruda realtà dei numeri sbugiarda ancora una volta il vice *premier* Di Maio, che ancora oggi ha l'ardire di dichiarare di poter garantire il blocco dell'aumento dell'IVA e di mantenere tutti gli impegni, ma anche Salvini e Giorgetti, che con spocchia considerano le clausole di salvaguardia sull'IVA solo un *escamotage* contabile: forse non se ne sono accorti, perché distratti e impegnati in altri giochi contabili, ma questa manovra ha annullato quel sistema. non saranno, ahimè, solo le vostre storie su Instagram, le *fake news* e la propaganda *social*, le foto coi gattini, o gli scatti che vi immortalano a volte con gli spacciatori puniti, e a volte con un *pathos* che fa il verso alle scene del documentario Olympia, ma le macerie che rimarranno dopo di voi. Le macerie di un Paese a cui state tagliando le gambe, a cui state cancellando prospettive di crescita, a cui state sottraendo la speranza e la fiducia. Un Paese che oggi viene riconsegnato ad un nuovo periodo di recessione, un inesorabile declino economico, ma anche culturale e solidale. Del vostro pessimo agire rimarrà la spocchia, la cattiveria e la doppia morale.

giorni precedenti in Commissione, ribadendo la nostra contrarierà ad una manovra finita peggio di come era nata, pensata esattamente al contrario di quelle che sono le reali esigenze del Paese. Fermatevi! BlackRock, l'altro giorno, ha detto chiaramente che gli investitori esteri non vogliono saperne più dei BTP italiani. Non si fidano più e non considerano più l'Italia come un Paese affidabile. In questo senso, l'immagine del *premier* Conte, ieri,

Fermatevi: ci state riportando nel *tunnel*. Signor Presidente, oggi è un giorno greve per l'Italia, perché abbiamo salutato un bravissimo ragazzo, un giornalista, Antonio Megalizzi.

Antonio era un amico e avrei voluto essere a Trento oggi, a salutarlo, ma penso che una giornata così richieda di salutarlo e che egli avrebbe voluto che fossi qui a dirvi le cose che sto per dire. *(Applausi dai una vita per la verità, per la democrazia e per l'Europa, con grandissimo rispetto per le istituzioni, è morto uscendo dall'istituzione del Parlamento europeo di Strasburgo e non avrebbe accettato minimamente quello che sta succedendo qui, oggi. Non parlo a un Governo che non ascolta, oggi non parlo nemmeno ad una maggioranza che non ha avuto la capacità di ascoltarci, ma parlo agli elettori che hanno votato questa maggioranza e dico loro che siamo solidali, che li capiamo e che capiamo la loro disillusione, perché adesso è oggettiva. È oggettiva l'incapacità di governare un Paese ed è oggettiva l'incapacità di scrivere una manovra che possa dipingere il futuro di questo Paese.

Non ci si comporta così nelle istituzioni. Volevano fare asse con i nuovi Paesi europei: abbiamo ascoltato Orban (l'ho ascoltato con le mie orecchie) e abbiamo ascoltato Kurz al congresso del Partito popolare europeo a Helsinki un mese fa. Sono stati i primi a dire che questa manovra non andava bene e che avrebbe contaminato in negativo tutta l'Europa in cui crediamo e che vogliamo migliorare. Volevate abolire la povertà e avete detto a tutti, in campagna elettorale, che c'erano risorse per 17 miliardi di euro, poi sono diventati nove, adesso probabilmente sono di cui un miliardo per i centri, che chissà quando partiranno, e due per il Rei, che ha introdotto il PD, e forse quattro miliardi, a residuo, per il reddito di cittadinanza. L'hanno già detto: 80 euro per forse 500.000 persone.

53.000 contratti a termine non rinnovati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Credevate talmente tanto nei contratti a tempo indeterminato che in questa manovra avete scritto che bloccate le assunzioni

E poi è un po' falsata questa cosa: con una mano si dà il reddito di cittadinanza, con l'altra si aumenta l'IVA per cui se uno fa un acquisto per rilanciare i consumi, si trova un'IVA altissima. una cosa inconcepibile. Volevate abbassare le tasse: accidenti! Le tasse sono altissime, tolti i crediti d'imposta sulla formazione e sugli investimenti, è raddoppiata perfino l'Ires (non se n'è accorto quasi nessuno) per gli enti non commerciali:

Volevate abrogare la Fornero. Ebbene, la Fornero c'è, è in vigore e il decreto che probabilmente cambierà qualcosa entrerà in vigore, forse, ad aprile e sarà una piccola finestra, di tre anni, per alcuni, con decurtazioni.

volevate la democrazia diretta, volevate essere ascoltati uno ad uno: è un diritto anche legittimo e lo capisco profondamente, ma qui - sappiatelo, cari elettori - non ascoltano nessuno e scrivono le cose in altri luoghi: in cinque, aiutati dagli altri cinque di Bruxelles, e qui le Commissioni non vedono niente. La Commissione bilancio, per cui siamo stati a disposizione per quindici giorni, non ha visto la manovra che arriverà domani. *(Applausi che questa imbarazzante situazione venisse trasmessa via *web,* perché tutti potessero vedere (ne avete fatto la bandiera per cinque anni), ma questa Bene, anzi malissimo. Questa cosa la voterete con la fiducia. Noi, la fiducia, davvero non possiamo darla. È veramente una questione di responsabilità, storica e sociale. Questa è una spirale antidemocratica. È una spirale veramente negativa per l'economia, ma anche per tutta la nostra società. Allora, lo dico e veramente lo voglio dire affinché resti agli atti: siamo di fronte a un *golpe* contro l'Italia e contro gli italiani. *(Applausi

esigenze alle quali la politica, evidentemente, negli ultimi vent'anni, non è riuscita a dare risposte esaustive e nemmeno sufficienti. Le istanze delle piccole imprese, delle partite IVA, dei professionisti: per questi soggetti abbiamo esteso il regime forfettario, innalzando la soglia per potervi accedere a un fatturato di 65.000 euro. Con questa estensione una platea molto più ampia di piccoli imprenditori potrà fruire non solo e non necessariamente di un risparmio fiscale, ma anche e soprattutto di una maggiore semplificazione tributaria, con l'esonero dagli studi di settore, dalla tenuta della contabilità, dalla dichiarazione IVA e da tutta una serie di adempimenti che condizionano negativamente l'attività economica. Si introduce anche una serie di interventi tutti finalizzati a venire incontro sempre alle esigenze delle imprese: dal taglio delle tariffe INAIL alla mini Ires, agli incentivi per chi assume giovani eccellenze, all'aumento della deducibilità dell'IMU fino al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Con quest'ultima misura andremo a saldare nel 2019 almeno il 50 per cento dei crediti che oggi le aziende vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Con la manovra verrà introdotto il reddito di cittadinanza. La narrazione sul reddito di cittadinanza che è passata negli ultimi mesi nella politica e, spesso, nell'informazione è fatta di frasi proferite - ahimè - anche da autorevoli esponenti di quello che dovrebbe essere il partito più rappresentativo della sinistra, quello che in teoria dovrebbe guardare alle esigenze dei più deboli. si sentono frasi quali «reddito di cittadinanza vuol dire dare i soldi alla gente perché non lavori» oppure «pagare la gente che sta sul divano» o ancora «il reddito di cittadinanza è un voto di scambio». Forse occorre rammentare a chi ha espresso tali considerazioni - secondo il mio modesto parere superficiali - che proprio pochi giorni fa, il 10 dicembre, si è celebrato il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, dove, all'articolo 25, è sancito che «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia». Il reddito di cittadinanza vuole dare una risposta a questa domanda, vuole introdurre nel nostro ordinamento siffatto principio. Per questo è necessario opporre a quelle superficiali narrazioni altre e diverse narrazioni, quelle che parlano di padri di famiglia, quarantenni, cinquantenni, che hanno perso il lavoro, per i quali si sono esaurite tutte le forme di protezione sociale esistenti e ora non hanno più nulla, nemmeno la possibilità di riqualificarsi, perché anche la formazione costa. Ci possono essere degli abusi, sicuramente; il rischio che si verifichino degli abusi è insito in ogni misura di *welfare*, così come anche nelle misure di agevolazione alle imprese; ma non per questo non dobbiamo introdurre quelle misure. Occorre adottare degli accorgimenti necessari per impedirli o ridurli al minimo. Ma questa risposta va data e andava data. L'introduzione del reddito di inclusione da parte del precedente Governo dimostra, in realtà, che l'importanza di introdurre un reddito minimo universale è stata in realtà anche se con una misura del tutto inconsistente, conseguenza, peraltro, di un dibattito che già noi del MoVimento 5 Stelle avviammo a partire dalla scorsa legislatura. Esistono anche altre misure espansive che potrebbero avere un effetto moltiplicatore più ampio sull'economia: gli investimenti, la realizzazione di opere pubbliche - anch'esse previste nella legge di bilancio, attraverso il fondo per la messa in sicurezza di strade - scuole e altri edifici nei piccoli Comuni. Si tratta di interventi con effetti macroeconomici forse più importanti nel medio e lungo termine. Ma alle persone che vivono in uno stato di indigenza e alle quali è stata levata ogni speranza di futuro non possiamo offrire solo visioni economiche articolate. Queste persone hanno bisogno di risposte immediate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E il reddito di cittadinanza è la nostra risposta immediata. Inoltre, tutte le risorse destinate a finanziare questa misura andranno a dare una spinta diretta e immediata ai consumi interni, contribuendo a rilanciare i settori economici dei beni alimentari e di prima necessità, che sono i principali settori produttivi e commerciali del nostro Paese.

che abbiamo dovuto ridurre il rapporto tra *deficit* e PIL e che la manovra è stata scritta da Juncker. Chi contesta sa bene che così non è. A tal proposito, vorrei concludere con una frase che ho letto qualche giorno fa in un articolo di un quotidiano che non si può dire stia proprio dalla nostra parte. L'autore dell'articolo ci contesta di aver comunicato troppo, ma conclude ammettendo che il risultato, in realtà, lo abbiamo davvero raggiunto e avremmo potuto benissimo pronunciare «Tutti ci assediavano e minacciavano di fare partire i mercati contro di noi e contro di voi. Abbiamo ceduto un po' per portare a casa il grosso. È la verità e tutti capirebbero». Presidente, è la verità e tutti capiranno. *(Applausi dal

su un testo che non c'è - seconda stella a destra - di una manovra di bilancio e del bilancio dello Stato che, alla luce del metodo con cui è stata costruita, fa coriandoli del nostro sistema democratico. Oggi facciamo polpette e ci mangiamo settanta anni di storia democratica di questo Paese. Per la prima volta, infatti, il Governo presenta la sua manovra senza passare per il Parlamento. Questa è una totale mancanza di rispetto delle procedure

le promesse elettorali di due movimenti distinti e distanti, con obiettivi politici distinti e distanti - il reddito di cittadinanza da una parte e quota 100 dall'altra

che, per realizzare un reddito di cittadinanza risicato e una quota 100 che disincentiva il pensionamento, si sono dovute mettere clausole di salvaguardia per 23 miliardi per il 2020 e per 29 miliardi per il 2021. ha un unico significato per il futuro del Paese: non ci sarà più flessibilità; non si potrà fare più niente, gli indirizzi e le scelte politiche saranno inibite. Con la spada di Damocle dell'IVA al 26,5 per cento nel 2021 torneremo al baratto.

chiunque verrà dopo come disinnescherà il prossimo debito e il prossimo *deficit* se il Paese viene buttato in recessione? Questo Governo dà soldi per finta alla gente perché, se da un lato elargisce uno spennacchiato reddito di cittadinanza, diminuito di altri 2 miliardi, dall'altro toglierà risorse ai cittadini facendo pagare loro il corrispettivo in imposte indirette. Lo stesso succederà con le pensioni e quota 100, con cui si cercherà comunque di disincentivare il pensionamento e i giovani rimarranno ancora fuori. Parlo ora di due argomenti a me cari: ambiente e cultura. Quanto al primo, fare finta di essere il Governo dell'economia circolare e poi mettere paletti e bloccare il sistema delle autorizzazioni degli impianti *end of waste,* al posto di emanare una semplice norma transitoria nelle more dell'applicazione della direttiva europea significa condannare un settore fondamentale come quello del riciclo dei rifiuti alla paralisi; di conseguenza ne risentirà l'ambiente e quindi il futuro, così ci ritroveremo con le strade e i magazzini pieni di rifiuti e tutto dovrà tornare agli inceneritori e ai termovalorizzatori da voi tanto vituperati. Gli spazi in discarica si stanno esaurendo; stanno aumentando vertiginosamente i costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese; si rischia il collasso se non si fanno ripartire gli impianti di riciclo e recupero e se non ne autorizziamo di nuovi al più presto. Inoltre - come ho ripetuto a più riprese - questo grido di allarme arriva da ogni contesto, da Legambiente a Confindustria passando per tutte le associazioni ecologiste e dalle stesse Regioni e Province in ogni parte d'Italia. L'altra questione la cultura e l'università. Fare finta di sostenere le università virtuose, consentendo loro di utilizzare i bilanci interni in attivo per procedere alle assunzioni del personale mancante e poi tagliare il fondo di finanziamento ordinario che è la principale fonte di entrata delle università italiane, bloccando nel contempo le assunzioni fino al 15 novembre 2019, come lo chiamate? Lo chiediamo al mondo universitario come lo chiamano? Per me è una beffa: o si toglie il blocco alle assunzioni o si elimina il taglio. In caso contrario si sta prendendo in giro la più importante istituzione culturale, l'università. Ma forse questo è molto lontano dai pensieri di molti di noi.

deve avere la vista lunga per guardare ben oltre la punta delle proprie scarpe, deve avere una visione di lungo respiro: questo fa la differenza. Noi non staremo certo ad assistere inerti e vi ricordiamo che le esperienze di Governo, se mal gestite, condannano. Quindi, state bene attenti a non scherzare con la buona fede dei cittadini e con tutta la classe produttiva italiana, che domani si accorgerà che nulla è contenuto in questa manovra che vada verso la crescita economica, verso l'incentivazione dell'impresa, verso la riduzione del cuneo fiscale e l'aumento dei posti di lavoro; che vada verso la semplificazione, quella vera e non certo quella farlocca che è stata presentata che comunque la Commissione europea - come hanno ricordato tanti colleghi prima di me - non promuoverà oggi la legge di bilancio, ma si riserva di decidere a fine gennaio e per questo siamo profondamente preoccupati, e non per non per noi ma per i nostri figli, di cui abbiamo la responsabilità. Chiedete a un genitore qualsiasi cosa sceglierebbe tra 80, 100, 780 euro al mese per sé, o la creazione delle condizioni perché il proprio figlio possa lavorare e garantirsi il futuro:

in attesa che l'astronave ci porti il testo definitivo della manovra, l'unica cosa che possiamo verificare con certezza è che il Governo nasce incendiario e finisce per essere pompiere. da quello che viene annunciato e da quello che abbiamo potuto verificare, finora si tratta di una manovra che è stretta tra le solite logiche ragionieristiche dell'Unione europea e la logica elettoralistica della maggioranza Grillo-leghista. È evidente - come è stato già detto da molti colleghi - che viene concessa una cambiale elettorale cadauno alle forze di maggioranza. Il Paese rimarrà sospeso fino al 1° aprile, che peraltro non è la data più seria del calendario - come tutti sappiamo in attesa di capire bene come funzioneranno queste due uniche misure, alle quali viene sacrificato tutto il resto dell'amministrazione

L'impostazione della manovra per noi è profondamente sbagliata. Noi di Fratelli d'Italia rimaniamo fermamente ancorati al programma con il quale ci siamo presentati agli elettori. Auspicavamo che ci fosse una scelta chiara e netta in favore delle imprese, del mondo della produzione, di tutti quegli italiani che, nonostante le mancanze del nostro Stato, continuano a fare il proprio dovere, a credere nella nostra Nazione, continuano e si ostinano a fare produzione e a creare lavoro. Certamente erano in attesa di scelte che fossero chiare e nette e che andassero nella direzione giusta di creare meno costo del lavoro in termini di tasse. Al contrario, mi sembra che ci si avvii a prevedere molte nuove tasse. Non c'è l'ombra della tassa piatta, che evidentemente è stata sacrificata rispetto a quelle che erano le principali fonti di propaganda elettorale; così come non viene mantenuta una serie di promesse, che a me piace chiamare impegni e che riguardano la vita

l'istruzione e la ricerca sono assolutamente insufficienti e continueranno a relegarci agli ultimi posti nella classifica delle nazioni che investono in futuro.

della scuola, personale docente e non docente, ai quali in campagna elettorale era stato promesso lo smantellamento della buona scuola. Invece, dopo tanti provvedimenti, arriviamo alla legge di bilancio e continuano ad essere disattese quelle promesse. Non ci sono misure significative

attraverso questa manovra, non vedranno mettere mano a quei lacci e lacciuoli che gli impediscono di liberare risorse e di fare scelte politiche di indirizzo sui territori.

Abbiamo problemi molto gravi di dissesto idrogeologico; abbiamo problemi molto importanti che riguardano le nostre infrastrutture e la sicurezza delle scuole. Mi sembra che i problemi che riguardano la quotidianità degli italiani e la tranquillità di tante famiglie vengano completamente ignorati anche nell'agenda politica. clamorosamente, una politica per il meridione d'Italia che è questione nazionale. Non si può pensare di dare attraverso il reddito di cittadinanza, il metadone di Stato, una risposta risolutiva al Mezzogiorno che ha sete di riscatto e deve avere reali possibilità per fare sviluppo attraverso quello che dovrebbe essere un serio piano di infrastrutturazione del territorio. Signori del Governo, serve veramente a poco, per non dire a nulla, avere un Ministro per il Sud senza avere una politica per il Mezzogiorno. anche rispetto a quello che era stato promesso all'impresa tipica italiana - penso ai balneari, penso al mondo del commercio, penso al mondo dei lavoratori autonomi si va verso una manovra che consegna il nulla assoluto e lascia assolutamente irrisolti i problemi e le gravi difficoltà che tali categorie vivono. Per tutti questi motivi non posso che concludere dicendo che la cacofonia aritmetica tra il e il 2,04 non farà altro che far sentire agli italiani la differenza sostanziale che c'è tra la parola cambiamento e la parola fallimento.

onestamente pensavo che essere qui a parlare della legge di bilancio dello Stato potesse essere per tutti noi l'occasione per parlare nel concreto

che sappiamo non avere nulla di quello che sarà il testo definitivo che ci verrà proposto domani. Discutiamo sostanzialmente immaginando i contenuti di una proposta che fisicamente non è ancora presente. Siamo qui a discutere dopo che la Camera ha votato la fiducia su un testo e probabilmente, fra qualche giorno, voterà un'altra fiducia su un testo diverso, in qualche misura mettendo in discussione la natura stessa dell'istituto della fiducia così come previsto dai Regolamenti parlamentari. Siamo qui a discutere dopo aver passato dei giorni in Commissione ad analizzare emendamenti; a sceglierne, tra tutti quelli presentati da parte dei vari Gruppi e segnalati, circa 500, che abbiamo commentato e discusso da un certo punto in avanti, sapendo che tutto il lavoro sarebbe stato totalmente virtuale, perché da altre parti qualcuno avrebbe scelto, senza alcun nesso con quella che è stata l'illustrazione degli stessi emendamenti in Commissione, quali inserire all'interno di un testo che sarebbe stato posto - lo sarà fra qualche ora - alla nostra fiducia, in un clima veramente

per dimostrare chi è più tosto, chi è più capace a comandare e a portare a segno un punto finale in una sorta di scommessa sulla pelle degli italiani. Sta di fatto che, nel concreto, ci è stato annunciato che sarebbe stata presentata una legge di bilancio che creava un *deficit* sul PIL del 2,4 per cento, quando tutti gli analisti ed economisti ci hanno detto, nelle stesse ore, che non era assolutamente immaginabile né sostenibile

dopo aver pagato questi maggiori interessi, ammontano a molte decine di miliardi le perdite sui patrimoni di tantissime società che li hanno visti svalutare. Sappiamo

Sappiamo che molti investitori stranieri hanno rinunciato a investire nel nostro Paese. Anche in questo caso, parliamo di qualche decina di miliardi di investimenti

gli altri parassiti e tutte le fitopatie esistenti. Abbiamo norme che intervengono a sostegno del settore della forestazione e della promozione dei suoi prodotti, ma poi sono state bocciate tutte le altre misure che vanno nella direzione di intervenire sui prodotti di montagna e tante altre proposte che abbiamo messo in campo.

tendenti ad affrontare il sostegno all'agricoltura sociale, alla tracciabilità dei prodotti e agli investimenti sui beni materiali, cui gran parte dell'agricoltura, anche se nominalmente, potrebbe accedere, ma, di fatto, così come è congeniata la norma non può farlo.

Avevamo poi proposto misure di sostegno alle filiere, che non sono state prese in considerazione. Avremmo voluto poter lavorare nel merito su tutti questi temi, confrontandoci con la maggioranza, consapevoli del nostro ruolo di minoranza, che

contributo è stato marginale, perché abbiamo presentato emendamenti che non sono mai stati votati e comunque non sappiamo se qualcosa di ciò che è stato presentato verrà in qualche misura preso in considerazione.

caso. Ci saremmo aspettati - forse ingenuamente - dalle forze politiche che si sono poste alla guida di un cambiamento nel rispetto delle istituzioni, e che nelle passate legislature ci hanno spiegato

centrata su misure di assistenzialismo e sulle pensioni; aumenta le imposte e le accise, riduce gli investimenti e il sostegno agli investimenti privati. Per tutte queste ragioni non solo siamo convinti

di ripresa che cominciava a dare segnali di sedimentazione e rafforzamento. È stata compromessa la fiducia nei confronti del Paese e soprattutto la possibilità di guardare con fiducia al futuro. Per tutti questi motivi riteniamo che sia stata e sia una grande occasione persa.

ragazze scandinave barbaramente sgozzate, dopo essere state rapite in Marocco da terroristi islamici, che hanno messo poi *online* il video terribile nel quale si vede mozzare la testa a una delle due ragazze. Questo fatto non può che non può che accrescere la nostra avversione al terrorismo e all'integralismo islamico ovunque si manifestino.

dove abbiamo potuto analizzare la legge di bilancio, evidentemente *sub specie* sanità. È stato possibile andare a fondo, e per me è stata un'occasione importante di incontrare tante associazioni di pazienti. La cosa che faccio più volentieri nella mia attività parlamentare è incontrare, se non direttamente i pazienti con i loro problemi immediati di salute, le associazioni che li rappresentano, rappresentano, le società scientifiche che in qualche modo se ne prendono cura, e insieme cercare di individuare quelle misure che possono migliorare la loro qualità di vita personale e qualità di vita anche in merito a quella che possiamo considerare la salute pubblica. È stato un lavoro interessante - ovviamente non abbiamo votato la manovra, ma abbiamo presentato una relazione di minoranza - un lavoro concreto sui contenuti, sulle possibilità di miglioramento. Per carità, non abbiamo votato quello che ci veniva proposto e loro non hanno votato nemmeno i nostri ordini del giorno. Ma l'obiettivo era sul pezzo: era a cercare di capire di che cosa ha bisogno oggi la nostra sanità e come noi possiamo, tutti insieme, dare risposta a una realtà che in fondo ci tocca tutti da vicino prima o poi. Devo dire che una piccola circostanza mi ha colpito molto e in qualche modo mi è sembrata perfino di buon auspicio.

a tutte quelle associazioni, a tutte quelle persone che dalla legge di bilancio aspettano risposte vere, risposte concrete. In alcuni casi sono risposte in termini economici; altre volte sono risposte in termini di semplificazione normativa; altre volte sono risposte che chiamano proprio in gioco norme concrete di cui il Paese ha bisogno per essere onesto davanti a un'altra affermazione di principio che ci caratterizza, che è quel famoso, amatissimo articolo 32 della Costituzione che considera la salute un diritto. Siamo l'unico Paese che considera la salute un diritto e che in questo senso considera norma costituzionale fondamentale la tutela di tale diritto. Facciamo molto in questo senso; non facciamo tutto ciò di cui c'è bisogno e, soprattutto, non lo facciamo per una serie di categorie di pazienti che meriterebbero maggiore attenzione da parte nostra e che dalla legge di bilancio aspettano risposte.

C'è stato un altro aspetto su cui mi sono soffermata: tutti noi sappiamo che la povertà è un'importante causa di malattia, è un elemento di comorbilità

tante patologie in questi anni, proprio grazie al contesto delle misure sociali. La povertà è importante come fattore fondamentale di salute. Non abbiamo creduto nemmeno per scherzo che si potesse abolire la povertà per legge, troppo facile. Noi crediamo a Gesù Bambino, a Roma crediamo perfino alla Befana, ma non crediamo che qualcuno possa venire raccontarci che la povertà si abolisce così, con colpo di bacchetta. Crediamo però - questo sì - che una legge di bilancio ben fatta riduca le disparità,

e che va a incidere sulla capacità di nutrirsi, sulla possibilità di curarsi, su quell'insieme di terapie non strettamente farmacologiche

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei cominciare questo mio intervento con una frase di *Kapuscinski**,* grande *reporter* e saggista polacco scomparso nel 2007: «È sempre il potere a provocare la rivoluzione. Non certo di proposito. Tuttavia il suo stile di vita e di governo finisce per diventare una vera e propria provocazione. Ciò avviene quando tra i personaggi dell'*élite* si instaurano il senso dell'impunità e la convinzione di poter fare qualunque cosa, di potersi permettere tutto». Quella che c'è stata il 4 marzo, colleghe e colleghi, è stata una rivoluzione. Una rivoluzione gentile, pacifica, fatta da milioni di cittadini che hanno deliberatamente scelto di dire basta a quel potere rappresentato dai vecchi partiti che per troppo tempo sono stati forti con i deboli e deboli con i forti. Questi cittadini hanno scelto noi, ci hanno dato una delle cose più preziose che esistano: la loro fiducia. Non intendiamo deluderli e questo disegno di legge di bilancio, la prima di tante, ne è la dimostrazione. In questi mesi, tra i banchi delle opposizioni, c'è stato chi ha avuto la faccia tosta di gridarci «Vergogna!». Beh, credo che a vergognarsi dovrebbero essere loro *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che - da competenti quali dicono di essere - ci hanno lasciato ci hanno lasciato un Paese con più di 5 milioni di persone in povertà assoluta, un Paese dove quasi la metà degli anziani non può permettersi nemmeno di accendere il riscaldamento nelle proprie case. Perciò di cosa dovremmo vergognarci? Del reddito di cittadinanza? All'articolo 1 la nostra amata Costituzione, quella che due anni fa qualcuno voleva stravolgere, recita che «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Ebbene, qualora non l'abbiate ancora capito - o peggio facciate finta - il reddito di cittadinanza è una misura per il lavoro, che permetterà a milioni di persone oggi escluse dal mercato e senza reddito di guardare al futuro con ottimismo. Dovremmo vergognarci di quota 100, con la quale iniziamo finalmente a superare la legge Fornero? Di aver disinnescato l'aumento dell'IVA nel 2019, una misura che mette al riparo i cittadini da un aumento del prelievo fiscale di oltre 12 miliardi? Di aver tagliato le pensioni d'oro e contemporaneamente aver alzato le minime? Degli 1,5 miliardi stanziati per i risparmiatori truffati dalle banche, quelli abbandonati da chi ci ha preceduti? Siate seri. Almeno per una volta, per favore, siate seri. Tra le pieghe di questa manovra ci sono provvedimenti che i cittadini attendevano da tempo immemore. Dopo una lunga confusione, per esempio, siamo riusciti a mettere un fondamentale punto fermo per i tanti professionisti sanitari che non si sono potuti iscrivere agli albi e, lavorando però in ambito sanitario, dopo la legge n. 3 del 2018 della Lorenzin, rischiavano di restare senza lavoro. I massofisioterapisti, per dirne una. Ecco, in questo caso - vi racconto rapidamente - chi fino al 1999 aveva frequentato dei corsi regionali abilitanti la professione ha ottenuto l'equipollenza con la laurea e la conseguente iscrizione all'albo dei fisioterapisti. Chi invece ha frequentato questi corsi, che continuavano a essere riconosciuti dalle Regioni, dopo il 1999 è rimasto fuori dall'albo e rischia adesso di non poter più lavorare. Con un emendamento inserito nel disegno di legge di bilancio, chi attualmente sta esercitando una professione sanitaria senza avere un titolo idoneo potrà continuare a farlo purché abbia svolto l'attività professionale per un determinato periodo negli ultimi dieci anni. Questo gli permetterà, infatti, di iscriversi in elenchi speciali ad esaurimento legati agli albi agli albi professionali. Naturalmente, non ci sarà un'equipollenza di titoli che consentano l'iscrizione agli albi, ma chi lavora potrà continuare a farlo: una notizia che aspettavano in molti e che oggi sono felice di poter dare. Non solo. Per gli enti territoriali - un altro capitolo che mi sta molto a cuore - istituiamo un fondo da 3 miliardi per il 2019, 3,4 per il 2020 e altri 2 per il 2021, che cresceranno fino a 3,2 miliardi annui nel periodo 2028-2033. Dal 2034 il fondo ripartirà con 1,5 miliardi annui. Andiamo ad aiutare Comuni, Province e Regioni su settori vitali come l'edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere a un miliardo di maggiori fondi derivante dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i Comuni virtuosi. Diamo ossigeno agli enti territoriali massacrati fino ad oggi dal Patto di stabilità interno e dal principio del pareggio di bilancio. In questo discorso, non possiamo certamente dimenticare il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nell'anticipazione ai Comuni in temporanea crisi di liquidità di risorse che potranno essere utilizzate per pagare i debiti nei confronti delle aziende. Finalmente da quest'Assemblea stanno uscendo provvedimenti che guardano ai reali bisogni dei cittadini, di tutti i cittadini. Finalmente si ricomincia a guardare alla politica e a chi occupa questi scranni con fiducia perché arrivano le risposte giuste.

mai nella storia repubblicana si è assistito a un atteggiamento così sprezzante nei confronti del Parlamento. Mi complimento con il sottosegretario

Eppure, vi è arrivato ieri il monito saggio del Capo dello Stato, che vi ha invitato a dialogare con il Parlamento, ad ascoltare le ragioni di chi, democraticamente, la pensa diversamente da voi. Capisco che siete in difficoltà. Partiti spavaldi contro l'Europa, minacciosamente spavaldi, ne avete dovuto accettare le indicazioni e le imposizioni; con arroganza infantile vi siete affacciati al balcone di Palazzo Chigi, annunciando al Paese la vostra rivoluzione economica, la vostra decrescita infelice. Ora da quale pulpito andrete a spiegare la vostra sconfitta e l'umiliazione cui avete portato l'Italia? Lo vedremo nei prossimi giorni. Il PIL con voi arretra, il debito pubblico aumenta e la crescita resterà ai blocchi di partenza. Insomma, approvate una legge di bilancio che renderà vulnerabile la nostra economia, che, faticosamente, iniziava a riprendersi. Poiché questo è e poiché questo hanno constatato e scritto i maggiori organi di stampa, avete iniziato a praticare un attacco vile alla libertà di stampa, nel tentativo di punire i giornali e i mezzi di informazione, che hanno raccontato i problemi del Governo e i suoi affanni strategici in economia. Vi siete chiesti come mai le categorie economiche e sociali del Paese sono in rivolta rispetto ai vostri provvedimenti? Le impazienze sociali si manifestano con intensità e con una piazza che, da Torino a Roma, si è messa le mani in tasca per non applaudirvi. La luna di miele col Paese sta comunque

Fornero, che era il *totem* da abbattere, rimane quasi inalterata, mentre la quota 100 avrà un periodo molto limitato per la sua applicazione. Avete solo innalzato un singolare, quanto ideologico, cartello dei no. No alla TAV, no alla TAP, no al buon senso, no agli investimenti seri per il Sud, che, con voi, ritorna ad un divario ineguagliabile

Volete che il Sud diventi una sorta di riserva indiana per anziani, senza agevolare attività economiche che possano rendere di qualità i servizi da fornire.

La vostra manovra, per me, ha un solo e fondamentale, elemento positivo: manda in ridicolo il vostro sovranismo alle vongole. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Avete dovuto cambiare linea. L'Europa brutta e cattiva - così dicevate con linguaggio sprezzante - vi è venuta incontro, ne avete dovuto riconoscere il primato e Conte lo ha capito. Intanto avete bruciato la nostra credibilità. Smettetela di giocare con finte riforme e pensate a come aiutare le imprese, pensate a come evitare di far fuggire gli investitori, pensate a ricostruire un tessuto di relazioni europee, dove l'Italia possa essere protagonista. Insomma, pensate. Oggi il vostro unico ossessivo pensiero è la lotta al passato. Ricordate che anche voi iniziate ad esserlo e l'incendio alle vostre bandiere sta lì a testimoniarlo. È una bugia dire che il Governo non sia arretrato. Il signor Presidente del Consiglio ha fatto una marcia indietro clamorosa, perché la sua manovra iniziale perché la sua manovra iniziale non reggeva alla prova dei fatti. Si preparano mesi difficili e purtroppo c'è il rischio della recessione. Il decreto dignità la sta anticipando sul fronte della disoccupazione. Fermatevi, per il bene del Paese, accettate il confronto. Avete detto che le opposizioni hanno presentato troppi emendamenti. Vi ricordo che dietro quegli emendamenti c'è il popolo, quel popolo che richiamate in ogni vostro discorso. PD).*Evidentemente non lo rispettate davvero, altrimenti avreste speso tempo a lavorare in Commissione e non a mortificare quanti avrebbero voluto confrontarsi

onorevoli colleghi, nell'introdurre alcune brevi considerazioni sul disegno di legge di bilancio che ci apprestiamo a votare, mi sia preliminarmente consentito rivolgere il mio personale apprezzamento - ma credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi del Gruppo del quale faccio parte, il Gruppo della Lega Salvini-Premier-PSd'Az (sia ben chiaro, questo è un aspetto importante della nostra denominazione

Aver evitato la procedura di infrazione senza rinunciare gli obiettivi che questa maggioranza si era data, primi tra tutti quota 100 e reddito di cittadinanza, corrisponde a un grande successo politico, checché ne dica L-SP-PSd'Az e M5S)*. Ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto,

Ma sul merito hanno sciorinato, come al solito, il libro dei sogni. Le opposizioni, durante la discussione della

Rappresenta la diversità tra chi reputa prioritari gli interessi italiani rispetto a chi è sempre stato succube della burocrazia comunitaria. Rappresenta la diversità tra chi vuole garantire serenità a chi ha lavorato per anni e, nel contempo, favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, rispetto a chi ha innalzato l'età pensionabile degli italiani alla più alta d'Europa. Rappresenta la diversità di chi vuole rimettere in moto il sistema Paese rispetto a chi ne ha rallentato la crescita. riferirmi a un argomento che mi sta particolarmente a cuore da rappresentante dell'associazionismo sportivo. C'è un argomento nel disegno di legge di bilancio che mi interessa e mi riferisco alla riforma dell'ordinamento sportivo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale: per anni ci siamo riferiti al nostro sistema sportivo incentrandolo tutto sulla figura del CONI, un'istituzione importante che sicuramente ha fatto un grande lavoro che ha, di fatto, supplito alle carenze dello Stato. Per tanti anni i nostri atleti sono andati in giro per il mondo, hanno rappresentato bene l'Italia e le hanno permesso di conseguire importanti successi che ne hanno migliorato l'immagine in giro per il mondo. Ma non c'è solo questo modo di intendere lo sport. C'è la necessità di sviluppare una cultura sportiva a gradi, che vada oltre gli aspetti competitivi e possa conferire allo sport una dimensione sociale e accentuarne i profili legati al benessere, al miglioramento della qualità della vita, all'educazione e alla prevenzione. Per anni lo Stato, in un eccesso di delega, ha attribuito al CONI le funzioni di un Ministero, senza che il CONI ne avesse né le risorse né le competenze. E se di colpe vogliamo parlare, queste non sono certo del CONI. È lo Stato che ha impedito l'affermazione sociale dello sport, trincerandosi dietro queste grandi vittorie e dietro le grandi affermazioni dei nostri atleti che hanno nascosto tutte le altre carenze. con questa manovra economica, lo Stato si riappropria della capacità di indirizzo in questa materia esercitandola direttamente. Non c'è alcun intento punitivo nei confronti del CONI, ma solo l'intento di ridistribuire ruoli e funzioni con chiarezza. Ci troviamo, quindi, di fronte a un passaggio di consegne tra un modello che ha esaurito la sua funzione e una concezione dello sport che mira ad esaltarne la sua funzione sociale. Ciò non deve farci dimenticare, però, quello che il CONI ha fatto nel corso degli anni, i risultati che ha ottenuto e il rispetto che merita questa istituzione. Al CONI va la nostra gratitudine e la nostra attenzione perché se l'è meritata nel corso degli anni. È stata la casa di tutti gli italiani che hanno fatto sport e continuerà a esserlo, in un contesto di rinnovamento che, di fatto, coinvolgerà tutto il sistema sportivo italiano. Ma noi, oggi, stiamo dando grandi impulsi

ogni forma di rispetto istituzionale che si dovrebbe a quest'Aula e ai senatori. Non abbiamo avuto la possibilità, il diritto e il dovere di esercitare quello che ci chiedono i cittadini, cioè di leggere, approfondire, intervenire, emendare ed arricchire la proposta di legge, in questo caso il disegno di legge di bilancio, che è la proposta di legge più importante. Ci ritroviamo qui vuoti, senza poter svolgere quello che ci chiedono i cittadini e quello che ci chiede la nostra carta costituzionale. Avete infranto ogni regola di rispetto verso le opposizioni, che si trovano oggi qui a parlare su un testo di legge che neppure conoscono. Avete giocato con l'Unione europea. Avete giocato e avete avuto cappotto. Avete mostrato i muscoli, ma io dico anche che i muscoli bisogna averli. O si hanno o non si hanno: se non si hanno, è meglio non giocare a *poker*, perché poi arriva il cappotto. consiglio davvero ai ministri Salvini e Di Maio qualche ora di palestra durante le festività, perché i muscoli o li hai, e allora li mostri, oppure non li hai ed allora è meglio lasciar perdere.

vedere; 1,823 miliardi le risorse che il Partito Democratico e quel Governo così terribile che ha distrutto il Paese aveva postato per la famiglia. Rispetto alla nostra cifra, -100 milioni.

Certo che ve li riconosciamo. Peccato che siano tutti investiti su iniziative proposte nella precedente legislatura. Avete semplicemente rinnovato quello che voi contestate in questa serata, niente di più. Sulla famiglia Sulla famiglia tanto evocata, io ricordo l'audizione del ministro Fontana, che ci ha davvero proposto un'agenda di cambiamento profonda, radicale, davvero stupefacente. E noi siamo rimasti allibiti da questa lungimiranza. Allora io vi domando, facendovi l'elenco, dove sono le proposte per la natalità? Dove sono le proposte per rilanciare i servizi per l'infanzia? Dove sono le proposte innovative per la conciliazione vita-lavoro? Dove Dove sono le proposte per il *welfare* aziendale? Ci vogliono queste proposte, se davvero la famiglia è il cuore del cambiamento. Noi non abbiamo visto nulla; avete riproposto

al quale vi invitiamo costantemente? Non farete altro - perché non c'è altra possibilità e non potete attivare i centri per l'impiego - che riproporre in versione vostra - ve lo concederemo cortesemente - il reddito di inclusione sociale. State riproponendo lo stesso meccanismo. Direte sicuramente che questo è il reddito di cittadinanza e che avete cancellato la povertà. Vi misureremo su questo, ma voi riproporrete lo stesso meccanismo e, guarda caso, nel dibattito pubblico ricompaiono i Comuni, scomparsi per mesi, ricompaiono le associazioni. Ancora una volta si tratta di una proposta farlocca,

prorogate ancora una volta il *turnover* e non fate altro che riproporre ciò che abbiamo già proposto. Lo state riproponendo. State vendendo fumo. Abbiamo discusso per tre giorni del decreto-legge concretezza, il nucleo della concretezza che avrebbe cambiato la pubblica amministrazione,

il grande assalto contro l'Europa, gli insulti contro i massimi rappresentanti della Commissione europea (che possono e devono bene essere criticati ma credo che gli quantomeno a livello internazionale, siano controproducenti) si sono risolti in una resa senza condizioni proprio a quella stessa Commissione europea Parlo di resa senza condizioni, anche se qualcuno dice che all'inizio la Commissione chiedeva un *deficit* inferiore al 2 2,4 per cento, con festeggiamenti al balcone, con la sconfitta della povertà e tutti gli altri annunci, annunci, con proclami di non muoversi di un millimetro, dicendo che delle lettere dell'Unione europea non interessava nulla; qualcuno ha sbattuto una scarpa sopra la lettera del commissario europeo;

l'attuale maggioranza ha sempre esecrato e additato al ludibrio quando lo facevano gli altri, cioè mettere le clausole di salvaguardia. La clausola di salvaguardia consiste nel fatto che voi colleghi della maggioranza state per votare (devo dire che avete poca alternativa, perché, così come a noi, anche a voi è impedito di avere qualunque tipo di influenza su questo disegno di legge, tranne di votare no, facoltà che vi resta) che vi resta) per scrivere nero su bianco che dal 1° gennaio 2020 aumentano pesantemente le accise sulla benzina. Ricordate il proclama di cancellarle al primo Consiglio dei ministri: in quell'occasione non si è fatto nulla, quando si arriva al sodo si mette nero su bianco che dal 2020 aumentano e nel frattempo restano assolutamente intatte, da quelle della guerra d'Etiopia a quella che si farà adesso dal 1° gennaio 2020 per il reddito di cittadinanza, che peraltro non c'è. Dunque, se non si interverrà, queste clausole di salvaguardia entreranno in vigore. Conosciamo bene le difficoltà che ci sono state quest'anno quando le clausole di salvaguardia, che l'attuale Governo e l'Italia ereditavano da quello precedente, erano 12 miliardi, ma in questo caso parliamo di 23 miliardi. Cioè per pagare i debiti ci si indebita, ma molto di più. È sano questo modo di amministrare lo Stato? Un padre di famiglia che facesse in questo modo, quanto pensate che duri? Quanto pensate che duri prima che non arrivino a pignorargli tutto il pignorabile? *(Applausi dal Gruppo

Tria è un uomo di poche parole, ma con quelle poche parole si spiega molto bene. Grazie al fatto che il reddito di cittadinanza ci sarà solo per nove mesi, supponendo che ci fosse dal 1° aprile - lo sottolineo ci sono 72 euro all'anno, dopo c'è qualche milione in più, ma i mesi del 2020 sono dodici. A parte il fatto che, prima di fare quella spesa, bisognerà trovare i 23 miliardi per coprire le clausole di salvaguardia, scendiamo a 62,76 euro al mese (sempre al posto dei 780 promessi). La sconfitta della povertà si ha dando 62 euro al mese a qualcuno.

Assumere la gente o promettere di assumerla dovrebbe far guadagnare consenso. Sì, però si assumono non prima della seconda metà di novembre dell'anno prossimo. Io immagino che i tanti che aspettano un posto un posto di lavoro diranno che è meglio novembre dell'anno prossimo piuttosto che mai. Vero. Ma cosa vuol dire assumerli dopo la metà di novembre? Vuol dire che non si paga neanche una mensilità nel corso del 2019 e dunque tutto si ribalta sul 2020; altra polvere sotto il tappeto, perché poi quelli saranno assunti, a meno che non si pensi di licenziarli il 2 gennaio del 2020. Insomma. è un atteggiamento gravemente irresponsabile. Contemporaneamente si bloccano una serie di lavori pubblici, quelli su cui si può puntare per il rilancio, e si fa tutto questo impedendo al Parlamento di lavorare. La Camera è stata fatta lavorare su un testo fasullo, mentre il Senato non può esprimere neanche un voto, se non quello di fiducia. Sapete a cosa serve il Parlamento? Non serve solo per fare le piazzate, non serve per controllare i costi del Parlamento stesso (perché altrimenti sarebbe un tantino inutile), ma serve a fare in modo che le misure, in particolare quelle economiche, vengano discusse alla luce del sole, in modo che ciascuno possa votarle una per una. Il fatto di farle scrivere a qualche funzionario di Palazzo Chigi o altrove è la garanzia di dare via libera a tante marchette e marchettine. E poi ci venite a parlare della fine della corruzione: qui si fanno quelle da miliardi, si fanno quelle da centinaia di milioni *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, perché, se si lascia il potere a qualche persona,

Tanto di questi funzionari non si conosce il nome. Si conosceranno solo i vostri nomi, che giustamente sono coperti dall'immunità, grazie all'articolo 68 della Costituzione; ma la vostra coscienza non è protetta dall'esecrazione che gli italiani avranno quando scopriranno i rovinosi effetti di queste misure.

«La Voce del Canavese», «La Voce di Mantova» sono venti tra i grandi giornali di tanti territori italiani che, per una norma cervellotica, caro Presidente, contenuta in questo maxiemendamento, saranno costretti a chiudere tra due o tre anni, a ridimensionare completamente la propria attività. Ho citato solo i quotidiani locali, ma le aziende interessate da questo provvedimento sono oltre 150, occupano migliaia di giornalisti, editano mensili e settimanali, senza citare l'indotto e la ricaduta sui territori. È una norma vigliacca, signor Presidente, che produrrà i suoi affetti tra dieci giorni, quando le programmazioni dei bilanci di previsione delle aziende sono ormai fatte.

il senatore Crimi tante volte, anche con l'aiuto di tante persone del MoVimento 5 Stelle, che hanno voluto mettersi a disposizione, ma che non sono riuscite purtroppo a impedire questo drammatico provvedimento. Una norma che il Presidente della Repubblica dovrebbe assolutamente bloccare, perché mette in discussione il pluralismo stesso dell'informazione, un principio cardine della nostra Costituzione. Una norma che non dovrebbe essere nella disponibilità di nessuna maggioranza e che mai e poi mai dovrebbe essere modificata con un maxiemendamento votato con una fiducia, senza nemmeno un passaggio vero in Parlamento. Ho voluto citare questi quotidiani locali senza calcolare, appunto, quanto verrà colpito l'indotto, le famiglie, le aziende. Questo perché il MoVimento 5 Stelle, fin dalla sua costituzione, ha voluto iniziare una campagna, attraverso Grillo, pensando che probabilmente questo finanziamento servisse ai grandi giornaloni di Stato come «la Repubblica», il «Corriere della sera» e «il Messaggero» che noi abbiamo da sempre combattuto. Invece, cari amici e cari senatori, oggi il MoVimento 5 Stelle, con questa norma, regala tra maggiori vendite e maggiori introiti pubblicitari, oltre 200 milioni di euro ai grandi giornali. Quelli che (sbagliando perché la stampa non si combatte eliminandola) volevano colpire i giornaloni gli servono invece su un piatto d'argento un regalo di Natale inaspettato. E, con il silenzio della Lega, riesce probabilmente ad alimentare quello che a molti di noi viene in mente e cioè questa idea di formazione delle piattaforme e dei *blog* tanto cari allo stesso Grillo e alla Casaleggio associati, che sono purtroppo i veri *leader* di questo Governo. Ecco, quello che avete combinato ha una ricaduta sociale drammatica e devastante sui territori e sulle province. Il MoVimento 5 stelle non brilla certo per il numero degli amministratori locali, è un movimento nuovo, e non sa che cosa significhi un quotidiano per i territori, non sa che cosa significhi per le province, caro Presidente, narrare quello che accade nei piccoli Comuni sperduti di montagna. I quotidiani, quelli locali, sono degli avamposti di libertà e di giustizia, danno la possibilità di conoscere questi territori. Voi li avete tolti, li state distruggendo sull'altare del mondialismo, sull'altare dei grandi giornaloni e di queste grandi testate *social* come Facebook e Google, che solo in parte, in realtà, solo in parte, in realtà, volete colpire con una *web tax*, un'idea alla quale, se aveste avuto l'umiltà di parlarne nelle Commissioni, avremmo sicuramente dato il nostro contributo.

Rimangono deserti migliaia di esercizi commerciali gestiti da imprenditori italiani. Lì si doveva colpire per cercare di reperire i fondi necessari ad una manovra che doveva essere, quella sì, veramente di cambiamento. E invece no, si colpiscono le eccellenze italiane, quindi gente che fa affari in Italia, che paga i propri dipendenti 700 euro al mese e che paga le tasse in paradisi fiscali viene tutelata; vengono invece tagliate le gambe ai veri imprenditori, a migliaia di giornalisti che hanno studiato per fare quel mestiere e che tutti i giorni ci mettono la faccia. Il Governo, il presidente Conte e il sottosegretario Crimi, invece di distruggere un sistema sano, virtuoso e strategico per tantissime province italiane, doveva pensare ad una norma che obbligasse questi giganti a restituire il dovuto agli editori, che li rendesse responsabili delle *fake news* che diffondono, che prevedesse per loro le stesse sanzioni e le stesse norme che hanno sempre regolato l'editoria.

Questa è la verità. Mi dicono che non ci siano precedenti al riguardo. Comunque, a prescindere da questo, già ieri il Presidente del Consiglio si è lasciato andare a un a un tentativo di ragionamento, dicendo che, in fin dei conti e per certi versi, il fatto che non ci sia un aumento della crescita e del PIL potrebbe potrebbe anche essere positivo, perché ci consente di fare maggior *deficit*. Forse ho capito male io, ma mi pare che oggi diverse agenzie di stampa abbiamo riportato

delle cose ipotetiche, ma nei fatti abbiamo visto - lo sviscereremo forse domani in modo più concreto - che non sono contingibili, urgenti e nemmeno spendibili.

E voi siete il Governo del cambiamento, il Governo del popolo: avete fatto i conti senza il popolo. Vi chiamate Governo del cambiamento e siete il Governo dei sostantivi: il decreto «sicurezza», il decreto «dignità», il decreto «concretezza». Siete un Governo di sostantivi ma senza sostanza, quella sostanza che avete cercato di mostrare anche nel recente

il paradigma che avete nella testa, voi del MoVimento 5 Stelle. Mi rivolgo a voi, che volete rappresentare il popolo e siete - di fatto - coloro i quali pensano in modo drammatico al popolo italiano e non al dramma del popolo italiano e alla povertà. Pensate che gli italiani siano un popolo di corrotti, questa è la verità.

non modificherà in alcun modo la storia dei discorsi parlamentari e non avrà di per sé impatto nel dibattito. Credo Credo che voi abbiate avuto un'occasione, che avete però sprecato. Penso ad un fatto piccolissimo e marginale, che pure è contenuto nella legge di bilancio: l'introduzione della cedolare secca

abbiamo anche una paternità. Il governo Berlusconi è stato infatti il primo Governo che nel 2011 ha introdotto questa misura, che ha consentito di risolvere un problema, anzi di diminuire l'area l'area dell'elusione fiscale, recuperando alle casse dello Stato circa un miliardo in poco più di sei anni. Parlo della cedolare per quanto riguarda le abitazioni. L'introduzione che voi fate oggi è invece assolutamente inefficace perché è prevista solamente per il 2019, solo per un anno,

lo è anche nell'introduzione di una misura che non poteva e non può che far bene alle casse del Paese e alle tasche degli italiani.

il vice *premier* Salvini, parlando proprio di situazioni legate alla fiscalità immobiliare, ha detto che avrebbero tolto l'IMU e le tasse sui negozi sfitti. Tutto questo non si è visto. Tutto questo non l'avete fatto. Tutto questo, cari amici della Lega, purtroppo, devo appuntarvelo, è stata una promessa annunciata, tradita Non si tratta di un ammontare straordinario di soldi, ma semplicemente di circa 170 milioni di euro l'anno, ampiamente recuperabili nel corso del tempo, ma con effetti benefici e di giustizia sociale. non credo che che, parlando del settore immobiliare, il Governo del cambiamento avrebbe dovuto cambiare la politica che è nata dal 2011 in poi. Mi spiace non sia presente in Aula il presidente Monti, ma è dal suo Governo e dall'idea secondo la quale l'Italia aveva la tassazione più bassa nel settore immobiliare che si è costruita la tassazione ed un carico vessatorio, quasi espropriativo e predatorio per le le abitazioni e per gli italiani. Vi ricordo che il 90 per cento degli italiani sono proprietari della loro abitazione ed è lì il fondamento della ricchezza. Non siete riusciti ad immaginare nemmeno come contrastare quella politica

siamo qui questa sera, a quest'ora, per difendere la dignità del Parlamento. Siamo qui a discutere di una manovra *bis*, diversa da quella che è stata approvata con la fiducia alla Camera pochi giorni fa, senza neanche avere in mano il testo del maxiemendamento su cui verrà posta la fiducia. Infatti, non essendo stata posta la fiducia, non sappiamo nulla di quello che eventualmente potrà essere recuperato di quanto discusso, mai votato, mai valutato, mai approfondito nella Commissione bilancio, che per una settimana

di una previsione concreta di quello che poteva essere accettato, accettabile, discusso, reale e concreto. Guardate, non lo dico solo per noi dell'opposizione, ma anche a beneficio di voi della maggioranza, perché questa roba qui sarà passata sopra la nostra testa, ma è passata anche sopra la vostra testa: perché così come noi l'abbiamo imparata oggi guardando i giornali, ve la siete letta anche voi sui giornali. Per un attimo Per un attimo avevo pensato: ma qual è il progetto? C'è un Ministro per la democrazia diretta, qui andate proprio diretti: non passate neanche dal Parlamento per fare le cose. È questa la democrazia diretta? nella scorsa legislatura avessimo fatto una cosa del genere, presidente Taverna, sottosegretario Santangelo (Cioffi, dove sei? Lucidi?), sareste lì nei banchi del Governo, non perché governavate, ma perché avreste occupato i banchi e gli scranni, per protestare con la massima forza che avreste potuto avere.

dai Gruppi* *PD e FI-BP).* Questo è il Parlamento che dovevate aprire come una scatoletta e oggi neanche la diretta televisiva! Non si può vedere cosa si fa qui; è vero: è roba che non si può vedere.

La verità è che questa manovra è un esercizio provvisorio *(Applausi dal Gruppo PD)*, perché non sta in piedi. È un esercizio provvisorio perché provvisoriamente oggi la votiamo, ma non avrà la forza di resistere a niente. Perché il Paese ha bisogno di altro, ha bisogno di un altro equilibrio composto di azioni che non sono minimamente contenute in questa manovra. Il Paese ha bisogno di investimenti, di favorire il lavoro attraverso gli investimenti,

delle condizioni in Europa. È chiaro che il Governo sovranista che si fa riscrivere le condizioni della manovra dall'Europa è un grande successo! Ma non voglio soffermarmi su questo. Voglio dire che, nel momento in cui riscrivete la manovra, dite due cose. La prima è che quella che avete approvato alla Camera era un grande falso in bilancio: il più grande falso in bilancio della storia, perché conteneva numeri che non era non sostenibili sotto nessun profilo, a cominciare dalla crescita attesa, crescita attesa, cui era collegata tutta una serie di aspetti che dovevano essere il motore della rinascita di questo Paese. Oggi ci rimettete delle cose che hanno talmente la forza di essere considerate probabili che bisogna aggiungere delle clausole di salvaguardia gigantesche, perché non c'è certezza di quello che ci scrivete dentro.

parliamo ormai di sette-otto anni fa. La Francia mi sembra che l'abbia fatto nel 2014 facendo slittare gli adeguamenti di sei mesi. Ebbene,

che per noi veramente manderà il Paese in difficoltà è perché prima ci sono stati un Governo e una maggioranza che hanno percorso la strada difficile e che hanno cercato di tenere sotto controllo il debito e di appostare quello che si poteva sugli investimenti e non sulla spesa corrente. Questo è il punto. Voi godete di questo vantaggio, di questa storia positiva del Paese e oggi, grazie a questo, potete fare questo esercizio provvisorio. Io spero - concludo con una battuta

Purtroppo la manovra del prossimo anno è già fatta, perché l'entità delle clausole di salvaguardia cui bisogna porre rimedio vale abbondantemente una nuova manovra. Questa, se riuscirà a stare in piedi, è una manovra che basta per due anni e sarà veramente un problema per il nostro Paese superare questo momento difficile.

la prima di questo Governo, intende rappresentare un importante e radicale cambiamento di paradigma rispetto alle politiche non condivisibili adottate negli ultimi anni,

hanno aumentato il debito pubblico oltre il 131 per cento del PIL, hanno accresciuto la disparità sociale e la povertà, hanno portato il Paese sull'orlo di una nuova recessione. Le politiche di bilancio proposte, purtroppo, hanno assecondato la cosiddetta trappola del debito, della quale l'Italia, tra i Paesi europei, risulta tra i più colpiti. Nel negativo quadro economico che è andato delineandosi, solo la Germania è riuscita, in questi difficili e complessi anni, a ridurre il *deficit*, portando il rapporto debito-PIL dall'81 al 65 Il crescente vortice del *deficit* è diretta conseguenza di un paradigma perverso, sposato e sostenuto inspiegabilmente e irresponsabilmente dalle autorità europee, che hanno considerato la sola stabilizzazione finanziaria e la conseguente riduzione del debito come la panacea di tutti i mali. Tale prospettiva, basata sulle politiche di *austerity*, si è rivelata però illusoria e ingannevole perché, oltre a essere stata disattesa dalla crescita del debito e del *deficit* sia strutturale che complessivo, ha finito per rallentare e oggi arrestare il rilancio economico dell'eurozona, così come la ripresa economica del nostro Paese, peraltro unico, tra i Paesi del Vecchio continente, a non aver raggiunto i livelli di crescita precrisi. In questi anni l'Italia ha perseguito indiscriminati tagli alla spesa pubblica, generalizzati blocchi del *turnover*, inspiegabili riduzione degli investimenti infrastrutturali nel capitale umano e nella ricerca; incomprensibili regole che hanno irrigidito, al di là di ogni buonsenso, il mercato degli appalti, trasferito, per ragioni incomprensibili, la titolarità del debito pubblico ai mercati finanziari internazionali, adottando, peraltro, perverse regole di collocazione - mi riferisco alle cosiddette aste marginali - che contribuiscono a collocare il debito al tasso più alto offerto dal mercato. Mi chiedo e vi chiedo come è stato possibile prefiggersi di ridurre il debito in un periodo - quello passato di una congiuntura internazionale favorevole e con un mercato dei tassi di interesse vicino allo zero. La realtà dimostra che abbiamo forse perso una grande occasione, ovvero di ammodernare l'assetto infrastrutturale, tecnologico e intellettuale del Paese. Abbiamo continuato a sostenere la spesa corrente improduttiva, finanziandola e incrementando il debito. I rendiconti degli anni 2016 e 2017 evidenziano, infatti, lo squilibrio che si è venuto ad accentuare tra la parte corrente e quella degli investimenti, vero motore della crescita di un Paese. Nel 2017, a fronte di una spesa corrente di 550 miliardi di euro, abbiamo impiegato in investimenti circa il 10 per cento Oggi, inoltre, ereditiamo un Paese con un rilevante tasso di disoccupazione, salito a oltre il 10 per cento, indietro sul piano tecnologico, con una elevata e diffusa povertà - oltre 5 milioni di persone - e soprattutto con un ciclo economico e finanziario non strutturalmente in equilibrio. È diventato pertanto necessario rompere questa nefasta trappola del debito, che oramai tiene prigionieri in molti Stati europei e minaccia la stabilità sociale della stessa Europa, come dimostrano i recenti fatti violenti accaduti in Francia e in Ungheria. Nell'ambito di questa nuova prospettiva, all'attuale Governo si deve il merito di aver proposto una manovra di bilancio diversa:

Una manovra da circa 32 miliardi di euro, molto superiore rispetto a quella da 27 e 28 miliardi di euro degli ultimi anni, che potrà contare su una serie di misure, quali, ad esempio, l'aumento degli investimenti infrastrutturali e gli investimenti nel capitale umano, attraverso l'introduzione del reddito di cittadinanza, lo sblocco del *turnover* - contenuto del decreto-legge concretezza - e l'abolizione finalmente della legge Fornero, con quota 100. Il rilancio delle infrastrutture sarà poi supportato da nuovi centri di progettazione centrali e decentrati, dallo svincolo degli avanzi di amministrazione degli enti locali e dalla riforma annunciata del codice degli appalti. Reddito di cittadinanza e quota 100 rappresentano per noi investimenti *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)* e non semplici costi monetari, perché mirano a riqualificare il Paese e ad alleviare la povertà, a ridurre la disoccupazione e a garantire la pace sociale. Concludo, ringraziando il Governo e le forze politiche che lo sostengono, perché hanno dimostrato responsabilità e fermezza: responsabilità per aver dialogato con l'Europa e scongiurato la procedura di infrazione; fermezza per non aver rinunciato a soddisfare gli obiettivi e le promesse fatte in campagna elettorale. PRESIDENTE. Senatore Turco, la invito Diversi saranno le insidie e i pericoli. Nonostante ciò si deve perseverare e andare avanti con forza. Questa legge di bilancio è quella voluta dai cittadini italiani.

Presidente, signor Sottosegretario, capisco che l'orario non agevola l'attenzione, ma, come hanno già detto i colleghi nel corso del dibattito, siamo di fronte ad una manovra che c'è e non c'è.

con riferimento al reddito di cittadinanza, sono stati gli interventi di Grillo e di Casaleggio, che, comprendendo la difficoltà in cui si trova la maggioranza, hanno pensato bene di dire «bravo» a Di Maio per essere riuscito a inserire il reddito di cittadinanza in mezzo a tutte queste queste difficoltà e a questi cattivoni dei giornali, con le opposizioni che strillano e tutto il mondo che va contro il Governo del cambiamento.

credo sia necessario esaminare questo fogliettino. Alcuni punti sono già stati spiegati dai miei colleghi. Ad esempio

ha spiegato chiaramente che la questione delle clausole di salvaguardia sull'IVA non solo sono un debito, ma di fatto - e non sto a insistere su questo concetto - si fa finta che abbiamo una specie di pozzo da cui attingere circa 20 miliardi di euro all'anno, e poi non si sa bene chi ci rimetterà.

le questioni del fatto e non fatto, che già abbiamo avuto il piacere di leggere, riguardano, ad esempio, la vicenda delle pensioni

di invalidità sarebbero non aumentate, ma rivalutate, e poi vi è una serie di scaglioni a seconda di quello che si può considerare più o meno ricco per decidere le indicizzazioni. Per recuperare poi un po' di soldi, non abbiamo il taglio delle pensioni d'oro (questo lo spiegheremo, come spiegheremo tutto il resto), ma abbiamo il solito vecchio sistema del del contributo di solidarietà che hanno utilizzato tutti i Governi di questo Paese, prevedendo una finestra temporale perché altrimenti arriva la mannaia della Corte costituzionale.

Mas. Tanto l'Europa l'IMU non la toglie, perché parte comunque dal presupposto, se ci andate a discutere, che ci deve massacrare per quello che riguarda gli immobili, che sono uno dei patrimoni più importanti nel Paese.

che lo aspetto a patollo, perché non ho ben compreso questa storia delle assunzioni da novembre e se per caso c'è una differenziazione tra le straordinarie e le ordinarie, per cui magari Salvini si fa le sue e qualcosa dai ricercatori mettete dentro; ma i magistrati sono assunzioni quindi la famosa mega-*task force* di magistrati che dovrebbero risolvere tutti i problemi dei tempi della giustizia sicuramente fino al primo di novembre non si può fare. Per com'è messa non si possono neanche assumere quelli che dovevano essere assunti prima. Questo è un punto rilevante per quanto mi riguarda, visto e considerato che già ci sono nel *web* le dichiarazioni di Bonafede sulle sue grandissime e straordinarie assunzioni.

Ha anche detto che qui non ce ne siamo accorti (ed è vero), ma guardate che fuori la CEI se n'è accorta e tanto. Oggi allora vi dà addosso «Avvenire» e vi dà addosso la CEI.

chiederei, e lo chiedo perché c'è una diversa concezione politica, al vice *premier* Salvini, che oggi ha deciso di fare il proclama per cui non voterebbe il bilancio dell'Unione europea per il problema dell'agricoltura:

Alla fine, se uno torna da Bruxelles con le pive nel sacco può anche tacere, che è un po' più dignitoso, quantomeno sui giornali e in televisione.

vorrei innanzitutto riportare alla realtà i toni di quest'Assemblea ringraziando i colleghi della 5a Commissione per il lavoro svolto Grazie fino alla fine in vita anche gli emendamenti non segnalati, tant'è vero che molti sono stati riammessi e discussi. Nonostante gli sforzi, la 5a Commissione non ha completato il suo lavoro, e di questo non posso che essere dispiaciuta, ma ha discusso ed approfondito tutte le proposte anche delle opposizioni. Ne è scaturito il quadro di un'Italia che ha bisogno di interventi urgenti in ogni settore, dalle infrastrutture agli enti locali, dalle imprese al sociale. E questa è una situazione che, indubbiamente e realmente, è stata ereditata dal passato. Cari colleghi dell'opposizione, capisco il gioco delle parti ma non si può puntare il dito su un Governo che non ha ancora approvato la sua prima manovra di bilancio! Come non si può puntare il dito su una Commissione che ha posticipato i suoi lavori nell'attesa di un esito. Cosa stavamo aspettando, se non l'esito di una intensa trattativa con l'Europa? Una Commissione europea che inizialmente ci voleva impiccare all'1,6 di *deficit*-PIL, permettendoci di fare una misera manovra inferiore ai 15 miliardi di euro!

Non ci sarebbero stati ulteriori spazi per altre misure. Invece, è stato giustamente rivendicato un 2,4 per cento e, dalla contrattazione è scaturito un 2,04 La legge di bilancio ha dovuto sì ridimensionarsi alla luce dei nuovi numeri, ma non si è di certo snaturata come qualcuno afferma. I capisaldi della manovra uscita dalla Camera rimangono rimangono inalterati: quota 100, con superamento della legge Fornero, e reddito di cittadinanza, una tassazione unica al 15 per cento con innalzamento del regime dei minimi a 65.000 euro, che vuole essere un inizio della *flat tax*. Rimane scongiurato l'aumento dell'IVA, problema provocato non certo da questo Governo. Poi ci sono tante altre misure. Penso al raddoppiamento della detassazione sull'IMU dei capannoni industriali. Penso alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisto di beni materiali strumentali strumentali e l'incremento occupazionale. Penso all'introduzione della cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali. Penso alla Formazione 4.0 che è stata recuperata. Penso al capitolo investimenti pubblici: sarà una sfida! Ci viene contestato di aver destinato poche risorse sui fondi dedicati ad investimenti ed infrastrutture. Ma è una questione che, essendo mia prima esperienza qui in Senato, mi ha lasciata sbalordita: cosa serve destinare risorse alle infrastrutture se poi le risorse stanziate non vengono ripartite nel giro di qualche mese? Bisogna essere poi in grado di permettere a questi fondi di convertirsi in nuove infrastrutture, in investimenti che trainino la crescita, lo sviluppo, l'occupazione! Non basta stanziare! Ed è questa la sfida cui faccio riferimento. Ed è quello che sta cercando di fare questa maggioranza: sbloccare le risorse esistenti. Il Governo sta cercando di fare il massimo con gli spazi finanziari frutto della contrattazione vincente con la Commissione europea.

Martin Luther King nel suo famoso e celebre discorso dell'agosto del 1963 pronunciò una delle sue frasi più celebri: «*I have a dream*». Sognava la fine della segregazione razziale. Anche noi, donne e uomini del MoVimento 5 Stelle, più modestamente avevamo e abbiamo un sogno, quello di far ritornare la politica al suo ruolo originario, non più un'occupazione del potere, non più una grigia e sorda mala gestione della cosa pubblica, ma al contrario un'attività nobile e alta, un sistema organizzato di ascolto delle esigenze e dei problemi dei cittadini e delle parti sociali, un complesso articolato di individui e istituzioni in grado di dare risposte concrete e di buonsenso alle imprese, ai professionisti, agli artigiani e alle persone, specie quelle che soffrono. Negli ultimi anni chi ha governato questo Paese e l'Europa ha dimenticato l'obiettivo alto che deve avere la politica; ha dimenticato i cittadini e le loro sofferenze e ha privilegiato i potentati economici, gli amici, le banche e le organizzazioni finanziarie. Dal 2011 sono state adottate insensate e assurde politiche di *austerity* che hanno acuito i problemi invece di risolverli. Ci era stato detto che l'austerità era necessaria, che avrebbe risanato e portato benefici nei conti pubblici, che il nostro debito sovrano sarebbe diminuito e che tutto ciò avrebbe favorito l'occupazione. Ci dissero che dovevamo fare alcuni sacrifici, ma che ne sarebbe valsa la pena.

In questo stesso lasso di tempo i nostri concittadini che si trovano sotto la soglia di povertà assoluta sono raddoppiati, arrivando a 5 milioni. La disoccupazione è aumentata, il precariato e il cattivo lavoro sono esplosi; la cosiddetta classe media è sparita. In compenso, si fa per dire, chi era ricco è diventato più ricco e chi era potente ha aumentato la sua posizione di forza e privilegio. Queste politiche economiche dissennate e assurde dettate dall'Europa e messe in pratica supinamente dei precedenti Governi hanno segnato un trasferimento di ricchezza da una massa enorme di cittadini a un ristretto numero di privilegiati. Questo tradimento del popolo italiano perpetrato dai Governi che ci hanno preceduto e questo disastro epocale saranno riportati nei libri di storia che i nostri figli e i nostri nipoti leggeranno nei prossimi decenni. Il Governo del cambiamento ha voluto invertire questa tendenza e ha presentato una manovra rivoluzionaria che assicurasse l'equità sociale e che evitasse in Italia le proteste di piazza come quelle dei *gilet* gialli in Francia perché per noi la stabilità finanziaria deve andare di pari passo con la stabilità e l'equità sociale. Vista la portata fortemente innovativa ed espansiva di questa manovra è stata necessaria qualche settimana affinché gli organismi europei ne comprendessero compiutamente i benefici effetti. Grazie al lavoro svolto dal Presidente del Consiglio abbiamo evitato la procedura di infrazione, che, tra l'altro, sarebbe stata riferita al debito pubblico del 2016 e del 2017 e, quindi, dei Governi Renzi e Gentiloni Silveri, i vostri Governi

(quindi sistematicamente) di sforare i limiti previsti dai trattati europei, come succederà nel 2019, pur di provare a placare i moti di piazza dei *gilet* gialli di cui parlavo prima. prima. Grazie alla bravura del nostro Governo abbiamo evitato la procedura di infrazione senza rinunciare minimamente ai capisaldi del contratto di Governo e del programma elettorale del MoVimento 5 Stelle, quindi senza rinunciare in alcun modo al reddito di cittadinanza, all'aumento delle pensioni minime di invalidità e alla quota 100 per il superamento della legge Fornero. Infatti, i contenuti dei provvedimenti, i tempi previsti, la platea dei beneficiari, gli importi che ad essi saranno erogati rimangono invariati rispetto alle previsioni e partiranno a fine marzo, esattamente come avevamo promesso. A chi oggi grida allo scandalo per le clausole di salvaguardia (che poi sono esattamente quelli che le hanno introdotte) diciamo di stare tranquilli: come abbiamo sterilizzato le clausole che voi avete messo per il 2019, allo stesso modo sterilizzeremo quelle per gli anni 2020-2021, perché con l'azione di Governo recupereremo miliardi di euro fino ad oggi sperperati per mantenere le vostre clientele e il potere, per favorire gli amici, per rimanere incollati a comode e ricche poltrone. La legge spazza corrotti, da noi fortemente voluta e approvata in tempi record, ci aiuterà molto in quest'opera. Nel prossimo triennio ci saranno investimenti per quasi 20,7 miliardi; inoltre abbiamo convinto l'Europa della necessità di mettere in atto un poderoso piano d'investimenti per la manutenzione del territorio, per scongiurare il dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza di ponti, strade e infrastrutture, perché vogliamo che tragedie come quella del ponte di Genova non accadono mai più. Abbiamo pensato anche agli artigiani e ai professionisti, alle piccole e medie imprese, adottando la *flat tax* del 15 per cento per ricavi fino a 65.000 euro, che quindi interesserà circa un milione di soggetti; dal 2020 ci sarà una *flat tax* del 20 per ricavi da 65.000 a 100.000 euro, quindi i beneficiari aumenteranno ancora di più. La manovra del popolo è equa, quindi ridurremo le pensioni d'oro a chi non ha versato i relativi contributi previdenziali, ma solo a questi ultimi Chi ha versato tutto non sarà ovviamente minimamente toccato e questa sarà la nostra ennesima misura temporanea di solidarietà nei confronti di chi sta peggio. Noi amiamo il nostro Paese, siamo orgogliosi di essere italiani e vogliamo che l'Italia torni ad essere un Paese guida per l'Europa e per il mondo; vogliamo che gli italiani vivano in un Paese più libero, più solidale, più giusto e più equo, un Paese di cui essere fieri. Tutta la nostra attività politica e di Governo è e sarà indirizzata unicamente a questi obiettivi *(Applausi

naturalmente punteggiata di tanti «me ne frego» e di *spread* mangiati a colazione; evidentemente questi *spread* sono andati di traverso visto che ieri il vice *premier* Salvini, che si faceva bello di queste frasi (tra l'altro neanche molto originali) non si è nemmeno presentato qui in Senato, nel momento in cui Conte è stato lasciato solo a raccontare il fallimento della politica economica del nostro Paese rispetto all'Europa

Faraone è a supporto, signor Presidente. Ma, dicevo, di espansivo in questa manovra cosa c'è? C'è la spesa corrente, C'è la spesa corrente, che è una spesa - lo dico tecnicamente - parassitaria e clientelare, che non ha nulla a che fare con le politiche espansive che

Ebbene, di tutto questo non c'è cenno, così come non c'è cenno per nulla della *flat tax*, questa grande manovra voluta soprattutto dalla Lega, che pensava a un'unica aliquota per

promessa non la vedremo né ora, né mai. Signor Presidente, vorrei concentrarmi molto velocemente su alcune questioni che sono state toccate solo marginalmente questa sera e che invece sono fondamentali: mi riferisco all'ambiente, al territorio e alle città. Ora, questi sono temi dei quali soprattutto i 5 Stelle si sono riempiti la bocca in campagna elettorale. Abbiamo appena concluso la Conferenza mondiale sul clima in Polonia, una conferenza annuale che si tiene ormai da venticinque anni, dopo il vertice di Rio del 1992. Ebbene, Ebbene, questa è la vera emergenza. Di tutte queste questioni all'interno di questa legge di bilancio non c'è assolutamente nulla. D'altro canto, è anche stato assolutamente rumoroso constatare come, mentre in Polonia il mondo parlava del proprio futuro e delle questioni più spinose, il Governo non abbia praticamente commentato; non si è letto nulla, nessuna posizione ufficiale o o ufficiosa sulle questioni fondamentali di cui hanno parlato e sulle decisioni politiche che sono state prese. Vede, signor Presidente, la questione dell'ambiente non è per soli esperti e non è una questione per gli ambientalisti da salotto, come qualcuno ha detto. È una questione centrale per noi e per i nostri figli e questo Governo se ne è totalmente dimenticato a partire dalla prima manovra nella quale doveva invece ricordarsene. D'altro canto, questo è del tutto coerente per un Governo che vede come azionista di maggioranza quella forza politica che, quasi esclusivamente (per fortuna dell'Europa), ha votato contro la ratifica del Trattato di Parigi, non più di due anni fa. Ed è del tutto evidente che quel disinteresse totale nei confronti del futuro nostro e dei nostri figli viene mantenuto nelle politiche nazionali, a partire da questo bilancio. Ciò non ci sorprende, anche perché questo Governo sta facendo sponda con il Trump degli Stati Uniti e con il Putin della Russia, che sono i due grandi ostacoli, grandi come un macigno,

del fatto che il mutamento ormai è strutturale e non contingente, ma manca anche qualsiasi politica di mitigazione, che è l'ABC e che viene ben prima dell'adattamento. Vede, signor Presidente, qui servirebbe un piano d'azione, dal punto di vista per esempio degli ecobonus innovativi; invece ci si limita a una mera proroga di tutto quello che era già stato stabilito dal Governo precedente. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Potrei leggere l'elenco degli ecobonus che sono stati messi a regime; qua semplicemente c'è una mera proroga. C'è la proroga sull'efficientamento energetico, sulla ristrutturazione edilizia e sull'acquisto di grandi elettrodomestici. Fine, punto. Questo avete fatto, al di là delle balle che avete raccontato in campagna elettorale. Nessuna fiscalità di vantaggio per chi produce beni riciclabili e riutilizzabili; nessuna misura per favorire la realizzazione dei centri per la riparazione e per il recupero; zero sull'economia circolare. Anzi, con un emendamento presentato da voi, che ha fatto incazzare sia gli ambientalisti che i produttori (complimenti, non è facile farlo), mi riferisco l'emendamento sull'*end of waste*, avete messo a rischio di chiusura e sospensione

perché ne abbiamo già discusso e se avete un po' di buona fede andate a vedere cosa avete combinato. Accenno solamente a quella genialata della centrale unica di progettazione che non sappiamo da quale mente possa essere uscita, dalla mente centralista di chi certamente non ha mai amministrato neanche un condominio del nostro Paese. pensare a livello nazionale ad una centrale unica di programmazione e di progettazione per gli appalti vuol dire non aver capito che in questo modo non si farà assolutamente nulla, che partiranno una serie di corsi e ricorsi per cui tutti gli investimenti locali, anche di manutenzione ordinaria, verranno bloccati. Questo accadrà. Zero sul diritto alla casa, zero sulla rigenerazione urbana, non c'è un intervento per la rigenerazione urbana delle nostre città. In generale, zero sulle città e sulle periferie, zero sulla mobilità sostenibile, sulle infrastrutture, sulle s*mart city*, sulla tecnologia intelligente, zero sull'energia in particolare sulla sostenibilità ambientale, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla *green economy*. Chiudo, Presidente, dicendo zero su innovazione, qualità e sostenibilità. Voi 5 Stelle dovete fare i conti con queste promesse. siete riempiti la bocca e i documenti di queste promesse e non c'è nulla di tutto questo. Concludo, Presidente, dicendo che noi siamo molto rammaricati perché ci eravamo messi a disposizione per migliorare questo provvedimento. Avevamo presentato alcuni emendamenti sul tema dell'ambiente, delle città e del territorio, sulle aree interne, sulla demolizione degli immobili abusivi, sui fondi per la morosità inconsapevole e per la Protezione civile, per il ripristino dei boschi e degli arenili colpiti dalla distruzione ambientale di ottobre e di novembre, sui nuovi ecobonus, per esempio per la l'istituto sul fondo solidale per le famiglie vittime delle catastrofi naturali, il sisma *bonus* e gli incentivi alla rigenerazione urbana. Di tutto questo non c'è traccia perché non c'è stata minimamente la possibilità di parlarne. *(Applausi

quando il mio Gruppo mi ha chiesto di intervenire francamente stavo per non accettare perché non abbiamo assolutamente capito ancora cosa voteremo domani e questo è molto, molto grave. Pertanto ho cercato di

con gli SMS del nostro bravo presidente, senatore Pesco, ma francamente dopo questi SMS non succede assolutamente nulla: nessun voto, nessuna discussione, nessuna audizione, nessuna pubblicità.

non l'avrebbe autorizzato. A noi risulta che il presidente Alberti Casellati avesse autorizzato immediatamente la pubblicità dei lavori della Commissione bilancio, cosa che non è stata fatta. Avevamo chiesto l'audizione almeno dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Approviamo una legge di bilancio senza aver sentito cosa ne pensa l'Ufficio parlamentare di bilancio. È come se, in una società di capitali, l'assemblea dei soci votasse il bilancio senza leggere o ascoltare la relazione del collegio sindacale. Non si può.

Ci sono qui due colleghi, che, come me, fanno parte dell'Associazione italiana arbitri: il sottosegretario Santangelo e il senatore Castaldi. Il regolamento del giuoco del calcio è fatto di

fare. Fino a oggi, di tutte queste cose annunciate con grande prosopopea, non abbiamo visto assolutamente nulla. Nel merito di quello "straccio" che è passato in Commissione alcune cose sono però abbastanza chiare. È abbastanza chiaro che avete messo un'ipoteca almeno sulle prossime due leggi finanziarie (quelle del 2020 e 2021). Infatti, con le clausole di salvaguardia di 23 miliardi nel e 26 miliardi nel 2021 avete messo un'ipoteca grave per chi avrà la legittimazione di governare il Paese in quegli anni.

Noi vogliamo che tutti stiano meglio, non che diventiamo tutti un po' più poveri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. A noi piacerebbe che lo sviluppo del Paese passasse attraverso un innalzamento, laddove possibile, di tutti quanti i nostri concittadini. E non è con questi sei miliardi di euro miliardi di euro che si accontenta la base dei cinque milioni di poveri del nostro Paese. Li stiamo prendendo in giro - li state prendendo in giro - e giocare con la gente semplice può diventare gente semplice può diventare pericoloso. Vi siete affacciati al balcone. È un brutto segno per il nostro Paese, una pagina molto grigia e buia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non si gioca in questa maniera con la democrazia del nostro Paese. Chi si è affacciato al balcone ha fatto una brutta fine, ricordiamocelo sempre.

FI-BP)*. C'è qualcosa che, secondo me, non va. Avete bruciato 250 miliardi di capitalizzazione da quanto siete al governo.

Li avete tolti, non so quanto scientemente, ma sono stati tolti e sono stati bruciati. Avete detto che abolite la povertà. Io ho qualche dubbio perché, come diceva qualche collega, il risultato certo di oggi è che chi sta bene, sta sempre meglio, e chi sta male, sta sempre peggio. *(Applausi dal Gruppo azione. Avete detto che siete a favore del sistema connettivo e produttivo del nostro Paese e delle piccole medie imprese, quelle che rappresentano, specialmente nel Nord e nel Nord-Est, dal quale provengo io, il tessuto portante, la vecchia locomotiva del nostro Paese. Riducete il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, se non lo sapete, è quel sistema che permette ai piccoli e medi imprenditori di accedere al credito. Ciò vuol dire che il piccolo artigiano, il piccolo agricoltore e il piccolo imprenditore non possono accedere con questi fondi di garanzia al credito; un credito che costa sempre di più grazie alle manovre che avete fatto voi. La mancanza di accesso al credito nel nostro Paese è sempre più

Signor Presidente, colleghi e colleghe sono orgogliosa di discutere oggi di una manovra che finalmente mette in campo tutta una serie di risposte che il Paese attendeva da troppi anni; una manovra che ha deciso di investire innanzitutto sulle persone, quelle stesse persone da cui in questi anni sono giunte istanze sociali del tutto inascoltate da chi ci ha preceduto. Faccio sommessamente notare che mentre discutiamo la legge di bilancio, diverse esigenze sociali stanno esplodendo sotto i nostri occhi in altri Paesi europei, come in Francia. La legge ha il pregio di aver intercettato prima e meglio di altri queste esigenze, approfittando di misure ad altissimo impatto sociale come il reddito di cittadinanza, quota cento, aumento delle pensioni minime e i risarcimenti per i risparmiatori truffati dalle banche. La risoluzione e l'azzeramento delle ormai famose quattro banche, che ha ricordato nel suo intervento il collega Lannutti ha colpito in maniera consistente anche l'economia ed i cittadini del mio territorio, le Marche. Il fallimento di Banca Marche ha provocato l'azzeramento dei risparmi di una vita per migliaia di persone in una triste e cupa domenica pomeriggio di novembre del 2015. Permettetemi di portarmi questa testimonianza, in quanto ho ascoltato e visto da vicino le storie e le sofferenze di queste persone; piccoli azionisti e obbligazionisti, pensionati e piccoli artigiani che, investendo nella propria banca di paese, credevano di sostenere se stessi e l'economia del proprio territorio, non volevano speculare o arricchirsi, ma solo salvaguardare i propri risparmi per una vecchiaia serena e spensierata. Le attese di queste persone sono state deluse e tradite da uno Stato che non solo non li ha né tutelati né difesi, controllando in maniera doverosa e opportuna l'operato dei grandi *manager* e i bilanci delle banche, ma che di fatto li ha pugnalati alle spalle, azzerando con un decreto-legge tutti i loro risparmi, scaricando su di loro il fallimento degli istituti di credito e le ruberie di un'intera classe dirigente. Le tragiche storie dei risparmiatori, le loro lacrime e le loro proteste sono delle ferite ancora aperte. Colleghi, la maggioranza non si è solo limitata ad ascoltare queste persone, ma una volta arrivata al Governo ha considerato l'indennizzo e il rimborso di queste persone come un'impellenza e un obiettivo primario. Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle mantiene le promesse fatte in campagna elettorale, nonostante i vincoli europei e le ristrettezze di bilancio. Questo Governo ha stanziato 1,525 miliardi in tre anni per i truffati dalle banche del Centro Italia e delle banche venete, andrà a semplificare le procedure di rimborso attraverso i rimborsi diretti e, in via prioritaria, le famiglie con redditi più bassi. Includeremo gli obbligazionisti fino ad oggi esclusi dai rimborsi, a causa della complessità dei meccanismi di ristoro precedenti. Incrementeremo fino al 95 per cento il ristoro per gli obbligazionisti. Per quanto riguarda gli azionisti, finalmente potremo alleviare le loro ingiuste perdite patrimoniali attraverso un rimborso iniziale del 30 per cento, fino a 100.000 euro, per coprire la più vasta platea possibile. Una platea, però, che non contempla i grandi azionisti, i *manager*, i dirigenti e tutti coloro che avevano incarichi in consigli di amministrazione e di controllo, né tantomeno le fondazioni. Ma - ribadisco - il rimborso risarcisce solo i più deboli e gli indifesi. Ed eccoci qui a discutere e votare questa legge di bilancio, con la piena consapevolezza che, pur non cancellando totalmente i drammi e le ingiustizie passate, rappresenta la ferma volontà delle istituzioni di non permettere più che rimangano indifferenti e inermi di fronte a queste vicende. Mai più. Uno Stato e una politica di nuovo al proprio fianco, che tuteli i più deboli e che consideri la coesione sociale come la bussola della propria attività politica.

vorrei intervenire innanzitutto rispetto a quanto successo in 5a Commissione, anche in qualità di Vice Presidente. Sinceramente penso che

riprendere quanto già detto un'altra volta: che non funziona screditare l'intera categoria, l'intera Commissione; non ha senso. Si è verificata una situazione anomala? È vero. Avremmo voluto evitarla? Certamente. Avremmo di gran lunga preferito poter svolgere i lavori come quasi sempre è avvenuto, perché di intoppi - non come questo - ce ne sono stati sempre tanti. Ci sono state tante fiducie. Insomma, nessuno di noi è nato ieri e il più giovane qui ha quarant'anni, quindi non scandalizziamoci. Però questo lavoro è stato fatto. Soprattutto - ci tengo a dirlo perché fa parte anche questo del grande lavoro che, se vogliamo, è molto più faticoso di quello vero e proprio della Commissione - c'è stata l'interlocuzione con tutte le forze politiche presenti nella Commissione, alla presenza

vero che non manca mai che qualcuno, della minoranza e non dalla maggioranza, non gli faccia i complimenti proprio per la schiettezza, la chiarezza, la competenza con la quale interviene. interviene. Questo lo dico per tutte le persone che, sentendo qualche collega che dice che non abbiamo fatto niente, ci crede. E no, signori, siamo qui da settimane - ripeto - giorno e notte. E fa parte del nostro lavoro, non stiamo a fare gli eroi. Fa parte del nostro lavoro quando affrontiamo certi tipi di provvedimenti. C'è stata una discussione generale, tranquilli; c'è stata una fase di illustrazione degli emendamenti, che si è organizzata per argomenti e che si è conclusa prima, durante la quale il Governo è stato ad ascoltare e ha preso nota di tutto quanto è stato detto. Quindi queste fasi ci sono state. Avremmo potuto tranquillamente iniziare a votare come era stato anche preso in considerazione - tutte le proposte che sapevamo essere marginali e che sarebbero state sfoltite. Ci eravamo Ci eravamo detti tutti: sappiamo che la tempistica è molto stretta (perché lo sapevamo prima, certamente si è partiti in ritardo), quindi

iniziare a fare un'analisi delle ammissibilità e delle inammissibilità. Sono stati richiesti tanti ripescaggi, tante revisioni delle inammissibilità e questo è stato il lavoro dell'ultimo giorno e mezzo.

una voce che dica quello che è successo. Ripeto che in questo momento non parlo a nome né di una parte, né dell'altra, ma a difesa della Commissione. Purtroppo siamo arrivati a questo punto;